La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mattina, ha approvato modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 3 marzo del corrente anno. Oggi pomeriggio il Governo renderà comunicazioni sullo schema di decreto legislativo in materia di federalismo municipale. Seguirà il dibattito - per il quale si è proceduto alla ripartizione dei tempi tra i Gruppi - che proseguirà nella seduta antimeridiana di domani, fino alla votazione degli strumenti di indirizzo presentati. La votazione è prevista entro le ore 13,30 di domani. Nella seduta pomeridiana di domani, alle ore 16, il Ministro degli affari esteri renderà un'informativa sulla situazione in Libia. I Gruppi potranno intervenire per cinque minuti ciascuno. Il calendario di questa settimana prevede, inoltre, la discussione del disegno di legge sui prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, già approvato alla Camera dei deputati, nonché della mozione dei senatori Scanu ed altri sul poligono militare di Quirra. Giovedì pomeriggio si svolgeranno interrogazioni a risposta immediata con ripresa diretta televisiva. Il Ministro della salute risponderà a quesiti sul commissariamento della sanità in Abruzzo e sulla chiusura del reparto di malattie infettive dell'ospedale di Crotone. Le sedute della prossima settimana, a partire dal pomeriggio di martedì 1° marzo, saranno dedicate alla discussione di documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, nonché all'esame dei seguenti disegni di legge: squadre investigative sovranazionali; modifica delle circoscrizioni giudiziarie nella Regione Marche; nuova disciplina del prezzo dei libri; aumento del contributo a favore della biblioteca Regina Margherita; parità di accesso nei consigli di amministrazione delle società quotate (ove concluso in Commissione); ratifiche di accordi internazionali. Nella prossima Conferenza dei Capigruppo sarà calendarizzata la mozione a firma Vittoria Franco ed altri su donne e sistema dei media, insieme ad altre mozioni connesse. Onorevoli colleghi, avverto che, con lettera in data 17 febbraio 2011, il senatore Umberto Veronesi ha comunicato di rassegnare le proprie dimissioni dalla carica di senatore in seguito alla nomina a presidente del Consiglio direttivo dell'Agenzia per la sicurezza nucleare. Trattandosi di dimissioni originate da incompatibilità espressamente previste dalla legge, l'Assemblea non può che prenderne atto. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è autorizzata sin d'ora a convocarsi per procedere all'accertamento del senatore subentrante. Mi permetto di aggiungere - credo a nome di tutti voi - che spiace a questa Presidenza perdere un'autorevole figura del mondo della scienza e della ricerca come il professor Veronesi.

riassumo lo scopo e i principali contenuti della riforma. Lo schema di decreto sul federalismo fiscale municipale determina il passaggio epocale dalla finanza derivata alla finanza autonoma. Si tratta di un tassello fondamentale del percorso del federalismo fiscale, diretto a raddrizzare l'albero storto della finanza pubblica italiana. Fino ad ora ci siamo occupati del federalismo fiscale, quindi cerchiamo di raddrizzare la parte territoriale; in seguito, credo vi sarà la necessità di raddrizzare anche la parte storta a livello statale. Il federalismo serve ad avvicinare chi governa a chi è governato. In Italia si è decentrato il potere di spesa, ma non la responsabilità impositiva: questo ha favorito situazioni di inefficienza e non ha garantito un efficace controllo sugli sprechi, con conseguente danno per le tasche di tutti gli italiani. In un federalismo senza responsabilità, il cittadino non vede, paga e vota «al buio». Il quadro attuale della tassazione locale è caotico, essendo costituito da ben 18 fonti di gettito, che vanno dall'ICI alla «tassa sull'ombra», cui si aggiunge una zona grigia di prelievi di incerta natura (ad esempio, i canoni idrici), spesso oggetto di pronunce chiarificatrici della Corte costituzionale. Le finanze comunali, oltre a questa selva di tributi e gabelle, causa di spaventosi contenziosi e di pesanti oneri burocratici, si alimentano anche di trasferimenti statali e regionali, per parecchi miliardi di euro, assegnati in base alla stratificazione nel tempo del criterio della «spesa storica», che in Italia per ben 35 anni ha sistematicamente premiato gli enti inefficienti e penalizzato quelli virtuosi. Il risultato è l'antitesi di un serio federalismo, il cui presupposto sarebbe invece quello di riconoscere una reale autonomia e consentire al cittadino di giudicare, con il voto, l'amministrazione locale: per Tocqueville, infatti, la democrazia iniziava con la pubblicazione del bilancio sulla casa comunale. Lo scopo della riforma è quindi quello di determinare il passaggio dalla finanza derivata a quella autonoma, sostituendo oltre 11 miliardi di trasferimenti statali annui - assegnati in base al criterio irrazionale della spesa storica - con tributi propri e compartecipazioni. Vengono eliminate o accorpate ben 10 delle 18 attuali forme impositive. Le imposte locali devono diventare tracciabili. Si tratta di una tracciabilità aiutata dai fabbisogni *standard*, che indicheranno per ogni Comune la spesa opportuna per ciascuna delle funzioni fondamentali. Se prima un sindaco poteva facilmente aumentare l'addizionale IRPEF e il criterio della spesa storica non consentiva alcun controllo agli elettori, già da fine 2011 un sindaco non potrà facilmente aumentare l'addizionale comunale in presenza di una spesa esorbitante i nuovi fabbisogni *standard*, visibili da chiunque sul sito del Comune. Si permette così ai cittadini di esercitare il controllo democratico sui livelli di governo che sono più prossimi alla loro vita: il controllo esercitato nella sequenza «vedo-voto-pago». E, se non vedo, o se vedo ciò che non va bene, non lo voto. Si tratta del massimo risultato di responsabilizzazione ottenibile, senza reintrodurre l'imposizione sulla prima casa, respingendo quindi quelle proposte che miravano, in vari modi, a reintrodurla, anche surrettiziamente, o con formule complicatissime e destinate a rimanere incomprensibili al cittadino, o con espedienti che avrebbero determinato l'effetto contrario ad una responsabilizzazione dei livelli di governo locale.

che con una tassa sui servizi avrebbe determinato probabilmente un incremento della pressione fiscale, utilizzando fra l'altro un allegato applicativo quasi incomprensibile e di fatto inapplicabile e una tassazione sulla prima casa che questa maggioranza ha da tempo rifiutato sopprimendo l'ICI sulla prima casa. L'allegato all'emendamento presentato, che, in termini di trasparenza, rende semplice la famosa «formula Giarda»,

seconda, quella del cosiddetto terzo polo, avrebbe portato alla reintroduzione dell'ICI sulla prima casa (tra l'altro, credo che in una delle risoluzioni presentate questa tesi venga anche sostenuta da parte del maggior Gruppo di opposizione), seppur con una sua detraibilità dall'IRPEF, con una serie di conseguenti difficoltà: come ci si sarebbe comportati a fronte dei cosiddetti incapienti? Questo cosa voleva dire, che il beneficio dell'ICI sulla prima casa lo avrebbero avuto le fasce medio-alte e non quelle più basse? Ovvero, la detraibilità totale di un tributo proprio comunale avrebbe stimolato i Comuni ad incrementare al massimo l'ICI sulla prima casa, con conseguente danno alle finanze dello Stato, vista la sua detraibilità, e la conseguente deresponsabilizzazione dei livelli di governo locale. Più specificatamente, nel merito, lo schema del decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale e municipale prevede, in due fasi, il riassetto delle modalità di finanziamento dei Comuni, con la soppressione della maggior parte degli attuali trasferimenti statali (appunto, circa 11 miliardi di euro per i Comuni delle Regioni a statuto ordinario) e l'istituzione di autonome forme di entrata. In sintesi estrema, nella prima fase, corrispondente agli anni dal 2011 al 2013, è prevista la devoluzione ai Comuni, relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio: del 30 per cento del gettito derivante dalle imposte relative ai trasferimenti immobiliari; del gettito IRPEF relativo ai redditi fondiari (escluso il reddito agrario) e alle imposte di registro e di bollo sui contratti di locazione; di parte del gettito derivante dalla cedolare secca sugli affitti; di una compartecipazione al gettito IVA. Nella seconda fase, che parte nell'anno finanziario 2014, inoltre, saranno introdotte nell'ordinamento fiscale due nuove forme di tributi propri dei Comuni in sostituzione dei tributi esistenti: un'imposta municipale propria sulla proprietà immobiliare, destinata, ferma restando l'esenzione sulla prima casa, a ricomprendere l'attuale ICI, nonché l'IRPEF, con le proprie addizionali, relativa ai redditi fondiari derivanti da immobili non locati; un'imposta municipale secondaria, sull'occupazione di beni demaniali o del patrimonio indisponibile, anche ai fini pubblicitari. Resta ferma, anche a regime, la disciplina della cedolare secca Infondata - devo ripeterlo: infondata - è l'affermazione che il federalismo fiscale determinerà un aumento delle tasse locali. lo avremmo invece avuto se fossero stati approvati gli emendamenti presentati in Commissione dai Gruppi di opposizione. Non ho mai voluto citare nomi o numeri, che peraltro sono facilmente calcolabili e ricavabili, si dice che bisogna ridurre la pressione fiscale e per sostituire 11 miliardi di trasferimenti magari si propongono emendamenti per aumentarli per più di 20 miliardi, mi sembra che i conti non tornino proprio. Nessuna ulteriore imposizione viene introdotta per effetto del decreto. La realtà è un'altra: l'addizionale comunale all'IRPEF, di cui il decreto sul fisco comunale dispone

Lo stesso vale per l'imposta di scopo, anch'essa introdotta dalla legge finanziaria per il 2007, tassa che viene restituita se l'opera pubblica che è destinata a finanziare non viene iniziata entro due anni. L'introduzione dell'imposta di soggiorno non è da ascrivere al decreto sul fisco dei Comuni, ma è in realtà da ascrivere alla riforma costituzionale del 2001 che, modificando gli articoli 117 e 119 della Costituzione, ha di fatto abilitato ogni Regione a stabilirla. Lo prova la sentenza n. 102 del 2008, con cui la Corte costituzionale ha dovuto riconoscere la legittimità dell'imposta di soggiorno introdotta, peraltro a carico dei soli non sardi, dalla Regione Sardegna. Il decreto sul fisco municipale, disciplinando l'imposta di soggiorno, ha quindi un effetto calmierante delle potenzialità che in astratto la Costituzione assegna alle Regioni e che, in assenza del decreto statale, potrebbero intervenire con propria legge su quella base imponibile libera e stabilire, ciascuna a favore dei propri Comuni, un'imposta di soggiorno ben più pesante, perché magari rivolta ai non residenti nella Regione e quindi non pagata dai propri elettori. Il decreto sul fisco comunale invece riduce le imposte: l'imposizione sui redditi da affitto passa al 19 e al 21 per cento rispetto ad una aliquota che oggi può superare il 40 Le imposte complessive sui trasferimenti immobiliari vengono significativamente ridotte: un punto percentuale di aliquota, che corrisponde a una riduzione del 10 per cento per gli immobili non prima casa e di oltre il 30 per cento nei casi di immobili destinati a prima abitazione. L'aliquota dell'IMU (la nuova imposta municipale propria, che sostituisce ICI e IRPEF fondiaria) è un'aliquota di equilibrio rispetto alle imposte che accorpa: è quindi a saldo zero per la pressione fiscale complessiva. Il Comune ha infatti la possibilità di variare in aumento o in diminuzione dello 0,3 per cento l'aliquota dell'IMU. Se il Comune mantiene l'aliquota allo 0,76 per cento stabilito dal decreto ci sono importanti risparmi: ad esempio, per un bilocale tenuto sfitto in una grande città (65 metri quadrati, categoria catastale A/2 e rendita catastale di 672 euro), il risparmio fiscale va da un minimo di 138 a 312 euro all'anno, a seconda dello scaglione di reddito in cui rientra il proprietario. Nel caso lo stesso immobile sia affittato, con un canone di 800 euro al mese, grazie alla cedolare cento il proprietario risparmia da 162 a 1.794 euro all'anno. E anche l'inquilino ha un guadagno, perché non dovrà più subire l'adeguamento ISTAT del canone. È importante precisare che è nella facoltà del Comune prevedere la riduzione dell'IMU fino alla metà per gli immobili produttivi e quelli dei soggetti all'IRES. In questo caso, anche le imprese commerciali e tutti i soggetti all'imposta sul reddito delle società non hanno aggravio, anzi hanno un risparmio: per dirla chiara, rispetto alle false voci che parlavano di patrimoniale, se i comuni dovessero esercitare questa facoltà le imprese pagherebbero circa la metà di quello che pagano oggi. Il Comune è cioè libero di decidere se: far far pagare meno, rispetto all'attuale situazione, i proprietari di seconde case e qualcosa in più alle imprese o solo a certe categorie di imprese; far pagare uguale, come oggi, a tutti; far far pagare alle imprese circa la metà di quello che pagano oggi (usando la possibilità di dimezzare l'IMU); far pagare meno tutti, usando al massimo ribasso la facoltà di manovra sull'IMU, realizzando risparmi. In questo ventaglio di possibilità rimesse all'autonomia impositiva dei Comuni, si gioca la partita del federalismo fiscale, che in un quadro perlomeno di garantita invarianza della pressione fiscale complessiva avvicina i governanti ai governati, permettendo il controllo dei secondi sui primi in merito al *trade off* tra quanto si paga in imposte e i servizi che si ricevono. Un altro aspetto fondamentale della riforma è che i Comuni saranno responsabilizzati in modo nuovo ed efficace nella lotta all'evasione fiscale: avranno accesso all'anagrafe tributaria, al catasto elettronico e ad altre informazioni utili a fare emergere l'evasione sugli immobili; tratterranno, da subito, il 50 per cento dell'extragettito prodotto; con i risultati della lotta all'evasione, potranno costruire asili o scuole. Lo stesso vale per le «case fantasma» (gli immobili mai accatastati). Facciamo due esempi. Moltissimi immobili, in modo disinvolto, sono stati trasformati in prima abitazione grazie alle cosiddette assimilazioni, consentendo così al proprietario di non pagare le dovute tasse sulla seconda casa; un immobile così assimilato a prima casa che dovesse avere i contatori che girano per brevi periodi dell'anno tornerà ad essere seconda casa e quindi a pagare le relative imposte. Oppure, gli immobili che oggi dal punto di vista fiscale risultano sfitti, che dovessero invece risultare con i contatori in funzione tutto l'anno, dovranno essere oggetto di contratti di locazione generando entrate fiscali certe. Chiarita in questi termini, si comprende come si tratti di una riforma di sistema destinata a durare negli anni, ben al di là delle contingenze politiche. Per questo il Governo ha inteso assicurare nell'esercizio della delega un continuo dialogo con le autonomie e con tutte le forze politiche, accogliendo, nei limiti del possibile, richieste, suggerimenti, correzioni, di cui faccio veramente un ringraziamento sentito. del metodo del dialogo e del confronto in Parlamento nei rapporti con i Comuni. Nella riunione del Consiglio dei ministri del 9 febbraio scorso, il Governo ha deliberato la nuova trasmissione al Parlamento del testo con modificazioni dello schema del decreto legislativo sulla base dell'articolo 2, comma 4, della legge 5 maggio 2009, n. 42, unitamente alle proprie osservazioni in merito. Il testo dimostra che l'approccio del Governo nel corso dell'esame parlamentare dell'atto n. recante lo schema del decreto preliminarmente approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 4 agosto 2010, si è caratterizzato per la massima apertura nei riguardi dei positivi contributi via via proposti da ogni forza politica, di maggioranza come di opposizione. Il dibattito parlamentare è stato infatti ampio, approfondito e aperto, e ha visto l'accoglimento non soltanto di molte delle numerose proposte avanzate da esponenti dei Gruppi di opposizione, ma anche di molte istanze rappresentate dalle autonomie locali. L'esame parlamentare infatti è iniziato al termine del confronto nella sede della Conferenza unificata e si è protratto complessivamente dal 9 novembre 2010 fino al 3 febbraio 2011. Il termine per la conclusione dell'esame parlamentare già sarebbe scaduto il 28 gennaio scorso, a seguito della proroga di 20 giorni, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge n. 42 del 2009. Il Governo tuttavia ha liberamente deciso di soddisfare la richiesta avanzata, di assecondare un supplemento ulteriore di esame, pur avendo, in base alla delega, piena facoltà di procedere comunque alla deliberazione finale anche in assenza dei pareri parlamentari. L'esame parlamentare si è svolto sia in seno alle Commissioni indicate dalla citata legge n. 42, sia in seno ad altre cinque Commissioni parlamentari che hanno espresso altrettanti pareri favorevoli e trasmesso rilievi alla Commissione bicamerale. l'esame si è articolato attraverso 10 sedute, che si sono particolarmente intensificate nell'ultima e decisiva fase, per un totale di quasi 25 ore di dibattito. Si sono svolte inoltre 10 sedute della Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati, per un totale di quasi quattro ore e 11 sedute della Commissione programmazione economica, bilancio del Senato della Repubblica, per un totale di oltre sei ore. Infine, per quanto riguarda le altre Commissioni, si contano 37 sedute complessive, per un totale di quasi 11 ore di dibattito. Si sono svolte inoltre 21 audizioni di tecnici delle amministrazioni, docenti universitari ed altri esperti e rappresentanze particolarmente qualificate di interessi. A tali approfondimenti istruttori sono state dedicate complessivamente quasi nove ore. Da questo esame - che, come si vede, è stato assai lungo e approfondito - sono emerse numerose proposte di modificazione al testo dello schema del decreto. Il Governo ha ritenuto di scorgere spesso in essa contributi effettivamente migliorativi, al punto da accoglierle in gran parte, facendole proprie, nel corso dell'esame. Su questa base, il relatore in Commissione bicamerale, onorevole La Loggia, ha presentato una propria proposta di parere in versioni che via via recepivano le diverse proposte, fino al testo da ultimo depositato al termine della seduta della Commissione stessa del 2 febbraio scorso. Tali proposte di modificazione sono state elaborate in seno alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale per poi essere integralmente fatte proprie dalla Commissione programmazione economica, bilancio del Senato della Repubblica, il cui parere, reso la mattina del 3 febbraio 2011, è stato poi recepito nel testo deliberato dal Consiglio dei ministri nella riunione dello scorso 9 febbraio. Successivamente, al termine dell'esame in sede di Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, la proposta di parere del relatore, onorevole La Loggia, unica posta in votazione, è stata respinta. Infine, la Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati, sulla base dell'esito dell'esame nella Commissione bicamerale, ha convenuto unanimemente di soprassedere all'espressione del parere. Il frutto del dialogo e del confronto parlamentare è ulteriormente indicato nelle osservazioni che accompagnano il testo nuovamente trasmesso dal Governo al Parlamento. A tale proposito, vorrei sottolineare che dei complessivi 70 commi in cui si articola ora il decreto, che consta di 14 articoli, quelli comunque incisi da modifiche originate da proposte dei Gruppi parlamentari nella Commissione bicamerale, con forte prevalenza di quelli dell'opposizione, sono ben 12, e generalmente di gran rilievo. Addirittura 22 sono, comunque, i commi del tutto identici ai corrispondenti commi della proposta di parere alternativa depositata, da ultimo, lo scorso 1° febbraio dall'altro relatore, senatore Barbolini, in quanto recepivano il dibattito emerso in Commissione. L'importanza che il federalismo fiscale municipale avrà sulle relazioni tra le istituzioni coinvolte e sulla vita quotidiana dei cittadini ha suggerito al Governo l'adozione di un metodo concertato e connotato dalla massima disponibilità al dialogo, anche nei riguardi agli stessi Comuni. Oltre, dunque, al confronto nella sede delle Commissioni parlamentari, il Governo ha continuato ad avere un dialogo serrato con l'Associazione nazionale dei Comuni italiani, che si è concretizzato in non meno di 10 riunioni a livello tecnico e politico con le rappresentanze locali. Numerose proposte di modificazione, a cui i Comuni si sono dichiarati favorevoli, sono state fatte così proprie dal Governo e sono via via confluite nella proposta di parere del presidente La Loggia.

Vediamo ora i pilastri del federalismo fiscale e municipale. Le principali innovazioni rispetto al testo dello schema dello scorso agosto, sulle quali si è verificata una convergenza tra il Governo e la sua maggioranza in seno alle Commissioni, i Gruppi di opposizione e i Comuni, attengono pressoché a tutti i profili maggiormente significativi dell'impianto del federalismo fiscale municipale. In proposito, è bene sottolineare che l'intero sistema di federalismo fiscale che sta gradualmente prendendo forma, non soltanto sul versante municipale, si regge fondamentalmente su due pilastri. Il primo è il processo di fiscalizzazione, ossia di trasformazione della gran parte degli attuali flussi di finanza derivata in strumenti di autentica autonomia tributaria a disposizione degli enti territoriali nelle forme dei tributi propri, dei tributi propri derivati e delle compartecipazioni al gettito di tributi erariali e regionali. Ridefinire un sistema fiscale complesso e stratificato come quello italiano è anche un'ottima occasione per imprimere una svolta nel senso della semplificazione. sul federalismo municipale riduce a 10 ben 18 delle attuali forme impositive comunali. Il secondo pilastro è la garanzia della perequazione, necessaria per limitare, per i territori con minor capacità fiscale, le disparità che in tutti i sistemi di finanza decentrata risultano connesse all'esercizio dell'autonomia tributaria. Perché sia chiaro per tutti: il federalismo è fatto per unire e non per dividere il Paese. La perequazione è pensata come strumento necessario per garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali. L'aspetto rivoluzionario del federalismo fiscale è che si stabilisce, finalmente, che i flussi finanziari perequativi non avranno più, per ciascun ente territoriale destinatario, una consistenza ricavata dal criterio della spesa storica, paradossalmente sperequativo verso chi era stato maggiormente efficiente. Il passaggio al criterio virtuoso dei fabbisogni standard segnerà la fine delle gestioni finanziarie, talvolta dissennate, che sono a tutti note. Per ciascun ente si conoscerà l'entità della spesa pubblica necessaria per garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali e si potranno fornire modelli di gestione efficace ed efficiente. L'architrave del federalismo fiscale, sostenuto da questi pilastri, è, in ultima analisi, un sensibile rafforzamento del legame tra responsabilità finanziaria e responsabilità politica degli amministratori di ciascun livello di governo. Questo legame, peraltro, sarà rafforzato grazie a meccanismi premiali e sanzionatori previsti dal distinto decreto legislativo in corso d'esame. Passiamo dunque in rassegna, attraverso i criteri di analisi appena ricordati, le modificazioni al testo dello schema approvato lo scorso agosto accolte dal Governo. le principali modificazioni concernenti l'autonomia tributaria, il riferimento è innanzitutto alle modificazioni riferite alla fase transitoria. Si tratta, in primo luogo, dell'introduzione di una compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto, pari al 2 per cento del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché della previsione di modalità che consentano di rideterminare, concordemente con la Conferenza Stato-Città, le quote delle devoluzioni del gettito della compartecipazione all'IVA: quest'ultima precisazione è stata in particolare richiesta dall'ANCI e si inscrive in un modello collaborativo di relazioni finanziarie che il Governo intende valorizzare. La modificazione inoltre riprende al tempo stesso, sia una proposta emendativa avanzata dal senatore Baldassarri, sia quanto contenuto nella proposta di parere del senatore Barbolini. Barbolini. Si è provveduto poi ad estendere anche all'anno 2012 la garanzia per i Comuni dell'attribuzione di un ammontare di risorse pari ai trasferimenti soppressi, sulla base di precise richieste avanzate dall'ANCI. Sul versante dell'autonomia tariffaria, infine, si prevede ora - ancora su richiesta dell'ANCI - che, sino alla revisione della disciplina relativa ai prelievi pertinenti alla gestione dei rifiuti solidi urbani (che il Governo conta di predisporre quanto prima) continuino ad applicarsi i regolamenti comunali relativi, sia alla cosiddetta TARSU istituita nel 1993, sia alla tariffa di igiene ambientale, prevista dal cosiddetto decreto Ronchi del 1997. Resta inoltre ferma anche la facoltà per i Comuni di adottare la tariffa integrata ambientale istituita dall'articolo 238 del Testo unico dell'ambiente. modificazioni riferite sia alla fase transitoria che a quella a regime, alcune interessano la fiscalità riferita al patrimonio immobiliare sito nel territorio di ciascun Comune. Il testo originario prevedeva una compartecipazione statale al gettito dei tributi della fiscalità immobiliare municipale: essa è stata eliminata. Al suo posto si attribuirà ai Comuni una quota del gettito derivante dai tributi della fiscalità immobiliare municipale riferiti alle ipotesi di trasferimento (imposte di registro e di bollo, imposte ipotecaria e catastale non relativa agli atti soggetti ad imposta sul valore aggiunto, tributi speciali catastali e tasse ipotecarie). Inoltre, per rendere più certe e stabili sin da subito le disponibilità finanziarie dei Comuni, si è provveduto a determinare già nel decreto legislativo la quota del gettito a questi devoluta, derivante dall'applicazione della cedolare secca sugli affitti, fissata al 21,7 per cento per l'anno finanziario 2011 e al 21,6 per cento per i seguenti, e sempre suscettibile di rideterminazione, con la garanzia di modalità condivise con le Autonomie. Lo schema di decreto consente che, a partire dal 2014, il gettito della cedolare secca sugli affitti possa essere devoluto interamente ai Comuni, con corrispondente riduzione della quota di compartecipazione al gettito dei tributi per il caso di trasferimento immobiliare

la facoltà del locatore di chiedere l'adeguamento ISTAT del canone annuo o altri aggiornamenti previsti a qualsiasi titolo. In questo modo, anche l'inquilino avrà interesse alla regolarizzazione fiscale del rapporto giuridico che lo lega al locatore, così da rafforzare ulteriormente la lotta all'evasione. A garanzia dei Comuni, poi, e su loro esplicita richiesta, sono ora previste modalità che consentono di rideterminare concordemente con la Conferenza Stato-Città le quote delle devoluzioni del gettito della fiscalità immobiliare (articolo 2, e dell'imposta municipale propria (articolo 8, comma 5), mentre per quanto riguarda tutti i tributi devoluti ai Comuni è previsto che le variazioni annuali del gettito rimangano assoggettate al principio di territorialità e non determinino modificazioni delle quote del gettito oggetto delle anzidette devoluzioni. In questo modo, si garantisce che una dinamica positiva delle basi imponibili (che è ragionevole attendersi negli anni a venire, quando avremo lasciato alle nostre spalle la crisi economica e finanziaria) rimarrà a vantaggio dei Comuni. dei Comuni. Tra le maggiori novità introdotte durante l'esame parlamentare in ordine all'autonomia tributaria di entrambe le fasi (transitoria e a regime) poi la previsione della facoltà, per numerosi Comuni (per i capoluoghi di Provincia e quelli inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, ma anche per le unioni di Comuni) di istituire un'imposta di soggiorno. I turisti corrisponderanno tale imposta insieme al corrispettivo dovuto alla struttura ricettiva in cui alloggeranno in misura proporzionale al prezzo e fino ad un massimo di 5 euro per notte. Di particolare interesse è il vincolo, per i Comuni percettori, ad impiegare il gettito d'imposta di soggiorno per interventi in materia di turismo, di beni culturali ed ambientali locali e per relativi servizi pubblici locali.

Infine, è prevista una parziale sospensione del blocco dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, introdotto nel luglio 2008 a fini di coordinamento della finanza pubblica. i Comuni riacquistano la facoltà di introdurre o modificare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF. Tale sblocco (nei limiti dello 0,2 per cento annuo), è molto significativo non soltanto perché soddisfa

di riferire lo sblocco soltanto ai Comuni la cui addizionale IRPEF non sia già attestata su un'aliquota superiore allo 0,4 per cento, che corrisponde all'attuale media nazionale: ovvero, si dà la possibilità ai Comuni virtuosi di esercitare modificazioni riferite alla sola fase a regime, si tratta innanzitutto dell'eliminazione dal testo dello schema preliminare della compartecipazione statale al gettito d'imposta municipale propria municipale propria (sul possesso), nonché della natura facoltativa dell'imposta municipale secondaria. Inoltre, è stata eliminata dal paniere delle nuove entrate proprie comunali l'imposta sul trasferimento immobiliare, che era originariamente prevista come imposta autonoma nell'ambito dell'imposta municipale propria. Sempre in merito all'imposta municipale propria, su richiesta dei Comuni,

Si tratta di un'aliquota di equilibrio rispetto alle imposte che accorpa, e quindi non determina alcun aumento della pressione fiscale per il contribuente. Anzi, se il Comune mantiene un'aliquota allo 0,76 per cento si potrebbero conseguire, come si è già esposto in apertura, importanti risparmi. Il testo del decreto continua a prevedere la facoltà di modificazione dell'aliquota, praticabile con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. Prevede poi la facoltà, per ciascun Comune, di deliberare aumenti o diminuzioni dell'aliquota, fissati ora ad un massimo di 0,2 punti percentuali (per gli immobili locati) o di 0,3 punti percentuali (per gli altri). i Comuni potranno abbassare fino alla metà l'aliquota applicabile a tutte le imprese commerciali e a tutti i soggetti IRES, così da incentivare la localizzazione delle imprese nel proprio territorio. L'assetto così impartito all'imposta municipale propria, che è stato in buona parte condiviso dall'ANCI, coniuga certezza e flessibilità, valorizzando peraltro l'autonomia di ciascun Comune nel finanziamento delle politiche pubbliche che ciascuno di essi voglia determinare. Infine, per gli atti soggetti ad imposta di registro in caso di trasferimento immobiliare, è ora prevista l'esenzione dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie, con contestuale soppressione delle vigenti esenzioni ed agevolazioni. Passo ora alle principali modificazioni concernenti la perequazione secondo i fabbisogni standard. In merito al secondo pilastro, ovvero alla perequazione in base ai fabbisogni standard, con riferimento alla fase transitoria sono state perfezionate le modalità di ripartizione delle risorse delle risorse che confluiscono nel Fondo sperimentale di riequilibrio: è stato valorizzato il criterio demografico, con una garanzia in favore dei Comuni minori e la previsione di misure premiali in favore dei Comuni che che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali secondo la manovra finanziaria estiva 2010. Per la fase a regime, in accoglimento di una rilevante proposta modificativa avanzata dal maggior Gruppo di opposizione, è stata introdotta l'istituzione nel bilancio dello Stato di un fondo perequativo, con indicazione separata degli stanziamenti per i Comuni e degli stanziamenti per le Province, nonché, per quanto riguarda i Comuni, con articolazione in due componenti (funzioni fondamentali e funzioni non fondamentali). Le modalità di alimentazione e riparto saranno definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in conformità con l'articolo 13 della legge 5 Va ricordato che un più definito e dettagliato assetto del fondo perequativo per la fase a regime era stato esplicitamente richiesto dall'ANCI. alle principali modificazioni concernenti la responsabilizzazione degli amministratori locali. Con riferimento alle modifiche relative ai contrafforti innalzati per incrementare l'autonomia tributaria, nonché la fusione tra le responsabilità finanziaria e politica degli amministratori locali, ricordo che i Comuni saranno maggiormente integrati nell'azione di contrasto all'evasione fiscale. Pretendere che un efficace contrasto all'evasione fiscale possa essere perseguito soltanto con l'azione dello Stato è pura illusione. Non basta, infatti, che una parte del gettito evaso recuperato sia assegnata ai Comuni che si siano adoperati nella lotta all'evasione, ma occorre anche fornire alle comunità più vicine al cittadino - innanzitutto i Comuni - gli strumenti necessari perché possano contribuire fattivamente alla lotta all'evasione. A tal fine, il decreto prevede ora che il sistema informativo della fiscalità assicuri sempre l'interscambio dei dati relativi all'effettivo utilizzo degli immobili, con particolare riferimento alle risultanze catastali, alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, ai contratti di locazione e ai contratti di somministrazione delle cosiddette utenze domestiche. Gli episodi di collaborazione tra taluni Comuni e l'Agenzia delle entrate hanno già condotto a risultati eclatanti, portando alla luce, ad esempio, il caso di un soggetto che pur essendo proprietario di 8 immobili non presentava alcuna dichiarazione dei redditi. In ogni caso, vorrei ricordare, da una parte, che il decreto porta dal 33 al 50 per cento la quota assegnata fin da subito ai Comuni del gettito evaso e recuperato grazie anche alla loro collaborazione e, dall'altra, che, fin dalla prima versione del testo, si è assicurata a ciascun Comune l'attribuzione del maggior gettito derivante dall'accatastamento dei cosiddetti immobili-fantasma, ossia quegli immobili che, alla data di entrata in vigore del decreto, non saranno stati ancora denunziati al catasto. Ricordo che stiamo parlando di circa due milioni di immobili. Inoltre, il decreto prevede ora una nuova definizione, maggiormente rispettosa del dettato degli Statuti di autonomia delle Regioni a statuto speciale, dei limiti in cui il federalismo fiscale municipale, sia nella fase transitoria che in quella a regime, ha applicazione nei rispettivi territori. Esso prevede, infine, che, in ogni caso, dall'attuazione del federalismo fiscale non possa derivare, neanche nella fase transitoria, alcun aumento del prelievo fiscale complessivo a carico dei contribuenti. Il federalismo, infatti, è fatto per ridurre le tasse: punto.

al primo aspetto, il Governo preannuncia che dovrà essere assicurato il coerente allineamento dei termini previsti dallo schema di decreto rispetto ai successivi interventi del legislatore. Mi riferisco, in particolare, al differimento al 30 aprile 2011 - previsto dal decreto-legge 30 dicembre 2010, n. 225 (cosiddetto decreto milleproroghe) nel testo modificato dal Senato - del termine per gli adempimenti relativi alla presentazione delle dichiarazioni di immobili non registrati in catasto. Dovrà di conseguenza essere adeguato al 1° maggio 2011 il termine di decorrenza per l'applicazione delle connesse sanzioni (articolo 2, comma 12, dello schema di decreto legislativo). Inoltre, il Governo si impegna fin d'ora a garantire che la determinazione dei gettiti su base territoriale sia realizzata, con particolare riguardo all'IVA, secondo un progressivo adeguamento delle capacità amministrative e gestionali. Quanto ai tempi, non può essere trascurato un ulteriore elemento che riguarda l'entrata in vigore della riforma: i Comuni attendono da tempo il federalismo fiscale municipale e ne hanno bisogno per poter presentare i rispettivi bilanci preventivi relativi all'anno finanziario 2011. Il termine del 31 dicembre scorso previsto dal Testo unico degli enti locali è già stato prorogato, secondo le procedure previste, al 31 marzo 2011, ma è chiaro che è assolutamente necessario che le ulteriori proroghe che si rendessero necessarie, benché giuridicamente fattibili, siano evitate o comunque limitate. I Comuni devono avere certezza sia delle risorse disponibili sia dei relativi tempi. A questo fine, già nel maxiemendamento al decreto-legge cosiddetto milleproroghe di fine anno, si è reso necessario prevedere che entro il prossimo mese di marzo il Ministero dell'interno corrisponda ai Comuni delle Regioni ordinarie un acconto pari a quanto trasferito nel primo trimestre 2010 degli introiti che spetteranno loro sulla base del federalismo municipale.

nonché del parere della Giunta per il Regolamento espresso nella seduta del 7 giugno 2006, all'attribuzione del seggio resosi vacante nella regione Lombardia, a seguito delle dimissioni del senatore Umberto Veronesi, ha riscontrato, nella seduta odierna, che il candidato che segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo della lista alla quale apparteneva il predetto senatore è Francesco Monaco.

cioè quello della disponibilità di dati numerici sull'impatto finanziario di questo provvedimento. Non mi riferisco ai profili di copertura finanziaria, che pure abbiamo esaminato facendo osservazioni critiche nei modi che potranno essere ricavati dai resoconti della Commissione bilancio, ma mi riferisco all'impatto economico‑finanziario delle misure sulle quali siamo chiamati a pronunciarci: rispetto alle autonomie locali, in particolare ai Comuni, ma anche rispetto alla pressione fiscale. Abbiamo ascoltato alcune dichiarazioni del ministro Calderoli che ci lasciano alquanto perplessi, come quella secondo cui si produrrebbe con questo provvedimento una riduzione della pressione fiscale a carico delle imprese, quando invece nel provvedimento c'è scritto esattamente il contrario, cioè che l'aliquota della istituenda IMU

- che le variabili sottese ai principi di delega erano talmente tante e la complessità di produrre una simulazione, almeno

del sistema finanziario degli enti locali. Lo stesso Ministro dell'economia e delle finanze, signor Presidente, dopo aver ricordato - cito testualmente - che «Se la scelta è quella del costo standard», così come è, «è evidente che prima bisogna avere il costo standard» - disse correttamente il Ministro dell'economia e delle finanze «e poi calcolare il meccanismo finanziario di finanziamento». Sta di

nella fase di emanazione dei decreti attuativi del federalismo fiscale, vale a dire quella in cui ci troviamo ora, sarebbero stati prodotti tutti i dati necessari per comprendere le interrelazioni tra i vari provvedimenti, gli effetti finanziari e Anzi, disse che era già *in itinere* un lavoro di elaborazione dei dati tecnici, alcuni dei quali sono stati messi a disposizione dei colleghi della Bicamerale e anche di tutti i componenti delle Commissioni bilancio,

parziale elaborazione era stata fatta sull'ipotesi di introduzione della compartecipazione IRPEF; senonchè, come tutti sappiamo, la compartecipazione IRPEF è stata sostituita, anche su nostra proposta, con la compartecipazione IVA. A seguito di tale modifica, il vice presidente della Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale, l'onorevole Marco Causi,

e chiedeva espressamente di investire il Dipartimento delle finanze ed il COPAFF per formulare nuove previsioni ed effettuare nuovi calcoli sulla base di queste innovazioni. Mi riferisco alla compartecipazione IVA, ma non è il solo problema. innovazioni contenute nel testo oggi sottoposto al nostro esame rispetto a quello non licenziato dalla Commissione bicamerale per il federalismo fiscale riguarda proprio il tema della compartecipazione dell'IVA,

molto meglio di me i colleghi che hanno attivamente e proficuamente partecipato ai lavori di quella Commissione. Nel fare espresso riferimento alla compartecipazione IVA, si stabilisce di assumere a riferimento per la compartecipazione IVA il territorio su cui si è determinato il consumo cha ha dato luogo al prelievo. Ora, a prescindere dalla bontà di questa indicazione

la regola che sovrintende al pagamento dell'IVA è quella del domicilio fiscale del contribuente persona fisica o sede legale: si paga l'IVA dove si ha il domicilio fiscale. Ai fini della compartecipazione, ciò che rileva è il luogo del consumo. Ciò significa che il Governo, a prescindere dal merito, sta introducendo una norma che determinerà uno spostamento corposo di risorse finanziarie da un territorio all'altro, all'altro, seppur con riferimento ad uno solo degli elementi del federalismo, quello della compartecipazione: ma noi non sappiamo niente su questo. È vero che il problema è fortemente attenuato nella fase di avvio

a regime questo problema sarà molto importante e noi non abbiamo nessun dato, nessun elemento per fare un apprezzamento. Non ce l'abbiamo noi, non ce l'ha la maggioranza e non ce l'ha il Governo. Se, invece, il Governo ce l'ha, allora ci deve fornire questi dati.

riferimento la Provincia, mentre sappiamo che i dati sono disponibili su base regionale. In ogni caso, vedrà il Governo come fare questo calcolo complicatissimo di disaggregazione e riaggregazione Ciò che è certo è che per i Comuni italiani oggi non è chiaro, almeno a regime, quale sarà l'entità dei trasferimenti, come saranno i loro bilanci e così via.

nostro Paese. Mi sarei augurato che in questa lunga gestazione del decreto delegato sul federalismo municipale - lunga, perché ne conosciamo tutti l'*iter* travagliato - si fosse avuta la possibilità di avere dei dati previsionali.

Signor Presidente, signor Ministro, colleghe e colleghi, va innanzitutto ricordato che se ora siamo qui, per discutere la comunicazione del Governo sul decreto in materia di fisco municipale, ciò lo si deve al presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e al suo rigore istituzionale. Se fosse stato per il Governo, infatti, il decreto sul quale l'apposita Commissione parlamentare il 3 febbraio scorso ha respinto il parere favorevole, sarebbe già legge. Da parte nostra, che abbiamo votato contro il parere in Commissione, che nel corso della discussione abbiamo presentato precise proposte alternative come hanno fatto anche le altre opposizioni, ci saremmo aspettati che il Governo cogliesse l'occasione per cambiare il testo e per accogliere almeno parte delle osservazioni emerse nella discussione, le quali sono state fatte proprie anche da un largo schieramento di opinione pubblica. Che queste osservazioni siano fondate me lo fa credere il carattere insolitamente difensivo dell'intervento che abbiamo ascoltato or ora in quest'Aula da parte del ministro Calderoli. C'è infatti qualcosa di molto serio che ci preoccupa e che dovrebbe preoccupare il Governo almeno quanto noi. A causa principalmente di questo decreto, ma in verità anche per l'attuazione parziale e spesso distorta che almeno fin qui è stata fatta delle legge n. l'espressione «federalismo fiscale» viene ormai associata all'aumento delle tasse, alla riduzione delle risorse per i Comuni, al restringimento dei loro spazi di autonomia impositiva. Altro che «vedo, pago, voto», ministro Calderoli: qui la verità è che i cittadini pagheranno sempre di più e voteranno al buio, perché non c'è alcuna responsabilizzazione delle autonomie locali, anzi c'è persino una riduzione di quegli spazi di autonomia impositiva di cui finora hanno goduto e questo è un dato incontrovertibile. Noi crediamo nella necessità del federalismo fiscale e nella bontà della legge che insieme abbiamo contribuito ad elaborare, in quella che ormai appare l'unica parentesi di confronto autentico tra maggioranza e opposizioni in una legislatura per altro caratterizzata da uno scontro continuo e senza tregua. La legge n. 42 è una buona legge perché attua il federalismo della nostra Costituzione. Quello dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere riconosciuti su tutto il territorio nazionale, e non quello della territorialità del del prelievo fiscale, principio inizialmente sostenuto da PdL e Lega contro il quale ci siamo battuti con successo. Guarda caso finora non c'è alcuna traccia proprio della ricognizione dei livelli essenziali delle prestazioni a legislazione vigente; ciò vanifica anche l'individuazione dei costi e dei fabbisogni standard dei diversi servizi, poiché senza i livelli essenziali non sarà possibile fissare gli obiettivi di superamento della spesa storica, così uno dei cardini del federalismo fiscale, che è stato ricordato anche poco fa dal ministro Calderoli, resta totalmente inattuato. Un altro principio fondamentale della legge n. 42, introdotto su nostra proposta, è il patto di convergenza verso i livelli essenziali dei servizi, cioè la destinazione di almeno una parte delle risorse derivanti dal superamento della spesa storica all'innalzamento dell'offerta di servizi nelle zone più deprivate del Paese, a partire dal Mezzogiorno. Anche di questo, che doveva essere contenuto nella decisione di finanza pubblica e nella legge di stabilità, non c'è traccia. L'altro pilastro della legge n. 42 è il sistema di perequazione di Regioni ed enti locali. Esso stabilisce che per le funzioni fondamentali degli enti locali e per i livelli essenziali delle prestazioni per le Regioni, lo Stato provvede alla perequazione integrale sulla base dei costi e fabbisogni standard, mentre per le altre funzioni e prestazioni la perequazione avviene con l'obiettivo di ridurre le differenze di capacità fiscali tra i diversi territori. E anche questo è un principio del tutto assente dai provvedimenti attuativi finora adottati. Tutto questo avviene in un quadro nel quale i decreti attuativi già sottoposti all'esame della Commissione e quelli che lo stanno per essere presentano ulteriori e gravi lacune: manca il sistema finanziario per le città metropolitane; mancano le funzioni e il sistema finanziario per Roma capitale. Le norme previste nei prossimi decreti sulla perequazione infrastrutturale e sugli interventi speciali per ridurre le diseguaglianze territoriali ricalcano meramente il testo della legge delega, e risultano perciò inattuate. Inoltre, la legge 42 non è stata finora accompagnata dalla Carta delle autonomie locali, la quale giace nella Commissione affari costituzionali del Senato senza che Governo e maggioranza mostrino una autentica volontà di completarne l'*iter*. C'è quindi una ragione di preoccupazione generale sul percorso del federalismo fiscale che oggi vogliamo sottoporre all'attenzione dell'Aula e del Governo, in aggiunta alle nostre considerazioni critiche sul merito del decreto al nostro esame. Se non si corregge rapidamente la rotta, il federalismo fiscale in via di attuazione non sarà quello della legge n. Sarà un'operazione di pura facciata, con il rischio concreto di produrre complicazioni ulteriori nel già fitto ginepraio del nostro sistema tributario, con effetti di deresposabilizzazione dei livelli locali e di una dipendenza ancor maggiore dell'attuale dalla finanza centrale. Vado ora ad illustrare rapidamente, nei pochi minuti che mi rimangono, le ragioni di merito per le quali il nostro Gruppo ha espresso parere contrario nella Commissione per il federalismo fiscale, parere peraltro contenuto nella relazione presentata dall'altro relatore, il senatore Giuliano Barbolini, che raccoglieva l'opinione di tutte le opposizioni. Essa poteva essere il punto di riferimento per riscrivere il decreto, per tener conto delle diverse opinioni, ma purtroppo così non è stato. Comprendiamo che l'ANCI abbia espresso soddisfazione perché alcune sue richieste sono state accolte, ma anche l'ANCI non ha mai nascosto le sue riserve sull'impianto complessivo del decreto. In primo luogo, non c'è un autentico legame con il meccanismo della perequazione ed ho già spiegato le ragioni per cui questo è molto grave. nel decreto manca completamente ogni corrispondenza con il principio federalista in base al quale i contribuenti di un comune devono coincidere con i beneficiari dei servizi, affinché si innesti il circuito virtuoso di responsabilità e autonomia in cui noi crediamo fermamente. Il Governo ha respinto la nostra proposta di introduzione di una Imposta comunale sui servizi che era sostitutiva, non aggiuntiva, delle attuali imposte sui rifiuti e dell'addizionale comunale all'IRPEF, e che veniva pagata da tutti i residenti non in quanto proprietari degli immobili, ma in quanto residenti in un comune. Mi sorprende che il ministro Calderoli si faccia spaventare da una formula matematica, peraltro molto semplice, che valeva a dimostrare come si voleva commisurare quel contributo non solo alla superficie dell'immobile, ma anche alla composizione del nucleo familiare. La proposta del Governo prevede che l'IMU, che è il principale tributo comunale sia pagato pressoché esclusivamente dai possessori di seconde e terze case, in prevalenza non residenti e quindi che non votano per gli amministratori chiamati a decidere su quella imposta. Altro che "vedo, pago, voto" Si mettono le tasse su quelli che non risiedono in quel comune. In più quella aliquota è chiaramente sottodimensionata, come tutti, anche le associazioni di impresa, hanno sottolineato, anche a questo livello - ma noi riteniamo che aumenterà ancora - determinerà un aumento di pressione fiscale eccome, ministro Calderoli, soprattutto sulle imprese e sui lavoratori autonomi. Ciò avviene per effetto della facoltatività della riduzione di imposta fino al 50 per cento per gli immobili ad uso produttivo e commerciale, mentre sugli immobili locati tale riduzione è automatica. è automatica. Lo sblocco delle addizionali IRPEF e il contributo di soggiorno si tradurranno da facoltà in obbligo ad aumentare le tasse, perché vi è stato nel luglio 2010 un taglio di 2,5 miliardi di euro sulle finanze dei Comuni che determina una diminuzione di risorse e quindi un obbligo per i Comuni, se vogliono recuperare, di applicare l'addizionale IRPEF che finora era bloccata. il Governo ha voluto inserire in questo decreto la cosiddetta cedolare secca sugli affitti. Si tratta di una norma che noi abbiamo richiesto per tanti anni, ma abbiamo sempre accompagnato questa proposta con forti riduzioni per gli inquilini, perché solo se emerge il conflitto di interessi tra proprietario e inquilino l'obiettivo di fondo che si propone questa misura, e cioè quello di far emergere il largo sommerso che è qui presente, potrà essere raggiunto. Così non sarà, perché il provvedimento del Governo non prevede alcuna detrazione per gli inquilini e in più ci sarà un buco nel bilancio dello Stato, come dimostrato dai documenti dei Servizi studi di Camera e Senato che pervicacemente non si sono neanche voluti prendere in esame. Inoltre, manca qualunque certezza e garanzia per quanto riguarda il il mantenimento delle risorse a disposizione dei Comuni dopo il 2012; il Governo ha infatti respinto un apposito emendamento in questa direzione. Concludo, signora Presidente, dicendo che il nostro Gruppo chiede al Governo di fermarsi.

Si discuta del prossimo decreto, quello sulle Regioni sulle Province, e dopo si torni a discutere in Commissione per il federalismo fiscale, una volta che il Governo abbia preso in esame quelle ragionevoli proposte di modifica che avanzeremo nel corso della discussione e che servono ad una autentica e reale attuazione della legge n. 42. Si sappia che il Partito Democratico - lo dico al Governo sul federalismo fiscale, come ha detto anche recentemente il nostro segretario Pierluigi Bersani. Siamo pronti ad assumerci le nostre responsabilità e a collaborare, ma per attuare la legge n. 42 e non per fare altro, che è in contraddizione con essa e che serve solo ad alzare qualche bandierina in vista di una possibile campagna elettorale.

alla schiera dei federalisti. Considero il federalismo una deviazione nel percorso che ha accompagnato per decenni il dibattito politico sullo sviluppo delle autonomie locali.

ma citando un grande intellettuale laico, azionista, Guido Dorso, che, nel suo impareggiabile saggio del 1924, «La rivoluzione meridionale», spiegava come l'autonomismo fosse una dimensione politica che viene prima di ogni configurazione e di ogni articolazione istituzionale: prima del regionalismo, prima del regionalismo, del federalismo, addirittura del modello di organizzazione degli stessi Comuni. Non vi è dubbio che questo spirito autonomista vero quello che si incarna principalmente nella dimensione locale, nella espressione della vita comunale: il Comune come cellula vitale della nostra democrazia.

compiendo chissà come - ma vedremo che non è così - un passaggio epocale verso una forma diversa dalla spesa storica. Nel 1978, la spesa storica non fu altro che la fotografia di quello che era avvenuto negli enti locali. Con una manovra gigantesca, che, secondo calcoli attuariali, varrebbe circa 50 miliardi di euro, lo Stato ripulì la finanza locale di tutti i debiti che si erano andati assommando, assunse su di sé quel debito e liberò lo spazio all'intervento delle autonomie locali. Non dobbiamo fare interventi algidi. Cosa ha significato quella operazione nel 1978? Una grande operazione di equità e di giustizia. Io ho cominciato le scuole medie

perché si faceva, appunto, il doppio e il triplo turno. Con quella operazione, negli anni Settanta, i Comuni furono messi in condizione di costruire scuole e asili nido, di creare un servizio sociale più esteso, di costruire le basi del nostro *welfare*. Per questo, bisogna riconoscere che quella operazione deve essere assunta come uno dei grandi parametri con i quali il nostro Stato ha operato una trasformazione profonda. Questo sta a significare che i trasferimenti, la politica con la quale lo Stato organizza il finanziamento delle proprie autonomie locali, non sono da demonizzare. C'è stata un'illusione, non vorrei definirla una distorsione grave, con la quale il legislatore ha voluto cancellare, riformando il Titolo V, la politica dei trasferimenti. Noi oggi dobbiamo operare senza avere di fronte il modulo del trasferimento, perché questo è stato cancellato e, quindi, dobbiamo sostituirlo con la fiscalità. Stiamo tornando indietro, perché fino al 1978 (quindi, per circa

che senza trasferimenti tutte queste operazioni rocambolesche sono senza un parametro vero, e che non c'è più un parametro equità. Nella sostanza, avverrà Nella sostanza, avverrà quanto già avvenuto nel silenzio qualche mese fa, con l'operazione della restituzione

avvenuto perché, quando si tocca un punto nevralgico della finanza locale, ci si illude che sia soltanto un fatto tecnico, mentre improvvisamente si determinano cambiamenti molto profondi.

La famigerata contrattazione, o negoziazione, con i sindaci che vengono a Roma con il cappello in mano per chiedere risorse sarà esattamente ciò a cui noi assisteremo nei prossimi mesi, perché l'unico criterio che sopravviverà sarà il negoziato dell'ANCI, che sta già preparando la documentazione, con il Governo.

che questa sia una logica accettabile, perché non è rispettosa per le autonomie locali. Come diceva Giorgio La Pira, infatti, le istituzioni sono il vestito

parliamo di soldi che vanno a finanziare i servizi delle nostre comunità. Abbiamo scelto come parametro l'IVA, al posto dell'IRPEF e siamo stati anche noi dell'opposizione ad acconciarci a questa soluzione. È giusto però che ci fermiamo a riflettere: certo, ormai è cosa fatta, ma, nel momento in cui diciamo che l'IVA va ripartita su base capitaria, se è vero che è l'unico criterio che ci rimane, sempre discutendo di manovre che si fanno avendo poche leve in mano, perché quello che avevamo prima, vale a dire l'organizzazione razionale attraverso il trasferimento, non si può più fare. Ma se la distribuzione

Qual è il principio che presiede a questa logica di finanziamento? Qual è il modo con il quale rendiamo giustizia ai territori che sono più ricchi e a quelli che sono più poveri? Tutto questo lo facciamo

e lo ripeto ancora una volta - è che non siamo in grado neppure di attendere la definizione dei fabbisogni standard, e quindi quella dei costi standard, perché nel frattempo, cioè già da ora,

Innanzitutto, secondo noi è importante capire come in questa fase questa riforma costituisca uno dei punti essenziali della politica economica del nostro Governo, un punto imprescindibile, e penso che su questo almeno dovremmo trovare una comune

«Il Sole 24 ORE» ha stimato in ben 150 milioni di euro (una cifra enorme) il potenziale recuperabile facendo emergere il 30 per cento di affitti che, anche nella virtuosa Milano, paiono essere in nero.

Presidente, rappresentanti del Governo, vorrei partire da alcune affermazioni che ha fatto il collega Garavaglia e che mi hanno particolarmente colpito.

in molti campi della spesa pubblica: penso, ad esempio, alla mancata occasione di ragionare sull'abolizione delle Province o su altre questioni che riguardano i Ministeri, gli uffici centrali e periferici

quindi fuggiti dalla tentazione, che pure era forte rispetto alla prima bozza sul federalismo, di porci con un atteggiamento semplicemente negativo o contrario. Abbiamo presentato una nostra proposta e moltissimi emendamenti (100 dei quali sono stati approvati); abbiamo provato a smontare e rimontare l'impianto della legge delega e, in parte, ci siamo riusciti, introducendo elementi che secondo noi sono molto significativi:

aspettative delle parti più arretrate, in termini di sviluppo e di servizi, del nostro Paese. Si deve imboccare certamente la strada della responsabilità fiscale,

Un nuovo patto fiscale basato sull'autonomia, sul decentramento e sulla responsabilità delle comunità non si può riscrivere né spezzando il Paese, né negando l'autonomia dei territori e dei Comuni, riaffermando, al contrario, una logica fortemente centralistica,

Abbiamo detto che era necessario definire i LEA, senza i quali non si poteva completare il circuito virtuoso rispetto ai fabbisogni standard, agli obiettivi dei servizi e, infine, al giusto riequilibrio attraverso la perequazione: tutto ciò è stato inutile. Si profila oggi un percorso normativo, peraltro, molto confusionario, in cui alcuni passaggi giuridici appaiono discutibili, come la previsione di decreti attuativi che rimandano ad altri decreti attuativi

all'impatto finanziario di questa manovra, tema che è stato posto in Commissione bilancio da parte di tanti nostri colleghi: ricordo inoltre numerosi interventi del senatore Morando in quest'Aula e in Commissione e finanche in questa giornata da parte del senatore Legnini. le nostre richieste e i nostri suggerimenti rispetto a questioni fondamentali per l'assetto di una riforma compiuta sono stati elusi. Non ci sfugge la complessità della manovra né che l'attuazione del federalismo richiede di destrutturare e ristrutturare la finanza locale e la finanza centrale, la spesa pubblica e l'assetto delle funzioni e dell'ordinamento e siamo consapevoli che un lavoro così serio avrebbe meritato approfondimenti più puntuali: partire con il piede giusto e fare tutti i passi in modo armonico. Non è stato così: abbiamo assistito a strappi ed ad accelerazioni immotivate. Quello che ne viene fuori in questo provvedimento sui fabbisogni standard è molto lontano dalle ispirazioni della legge delega e del tutto privo di un chiaro meccanismo perequativo, che è stato il punto essenziale dei nostri emendamenti e del nostro sforzo di ridefinire la legge delega. Senza un meccanismo di perequazione chiaro e definito, anche se tecnicamente da migliorare in fase di attuazione, non si potrà parlare di federalismo, né di autonomia, né si potrà richiedere una responsabilità

dei Comuni e un prevedibile aumento della tassazione per i cittadini e per le imprese. Ma questo non è il costo che si deve necessariamente pagare per l'attuazione del federalismo, bensì il prezzo di manovre profondamente centraliste, antimeridionalistiche, congiunturali e non strutturali (ritorno ai temi sollevati dal collega Garavaglia) che in questi anni ha deciso questo Governo, tagliando due miliardi e mezzo di euro ai Comuni,

evitando di piantare bandiere che potrebbero rilevarsi malpiantate e contrarie allo spirito che la riforma invece richiede. Signora Presidente, signori membri del Governo, colleghi, come ampiamente dimostrato dal precedente dibattito alle Camere e dal successivo voto che è stato espresso, l'Italia dei valori non era e non è tuttora contraria al federalismo, che impone una maggiore responsabilità degli amministratori verso i cittadini, ma ritiene iniquo il decreto sul fisco municipale, perché di fatto aumenta le spese, innalza le tasse, lasciando ancora più ingovernabili gli enti locali e i piccoli Comuni che ne segnalano le iniquità. Questo schema di decreto legislativo innova profondamente il testo a suo tempo presentato alla Commissione parlamentare e recepisce diversi rilievi

Diamo atto al Governo, e soprattutto al ministro Calderoli, di aver fatto l'impossibile per recepire i dubbi e le osservazioni che sono state fatte dal Gruppo Italia dei Valori, ma non siamo forse riusciti a convincere sulle nuove iniquità sociali che potranno derivare da questo testo. Nel corso dell'esame del provvedimento in Commissione bicamerale, anche attraverso la presentazione di un articolato parere alternativo, il Gruppo Italia dei Valori ha analiticamente evidenziato le criticità di ordine costituzionale e normativo, sia dello schema di decreto originario che delle proposte modificative. Si sono dimostrate le criticità del provvedimento e, nonostante le diverse modificazioni, si è dimostrato come i principi condivisi dal Gruppo Italia dei Valori in occasione dell'approvazione della legge delega n. 42 del 2009 si siano di fatto dissolti sotto il profilo formale e sostanziale. Trattandosi di fisco municipale, va sottolineato che la situazione economico-finanziaria degli enti locali versa in una situazione di estrema criticità, derivante dai rigidi vincoli del Patto di stabilità interno nonché, soprattutto, dalle ingentissime decurtazioni dei trasferimenti erariali messi recentemente in atto da numerosi provvedimenti di carattere normativo, tali da compromettere in alcuni casi l'erogazione di servizi essenziali per i cittadini. La sconfessione della legge n. 42 - su cui il nostro Gruppo ha in maniera convinta votato a favore - si attesta principalmente e sinteticamente su 3 rilevantissimi profili. la negazione del principio della maggiore responsabilizzazione economico-gestionale degli amministratori locali, l'autonomia tributaria riservata ai Comuni per tassare i non residenti, la tassa di soggiorno:

Il germe dell'indeterminatezza che infettava il precedente decreto legislativo sui fabbisogni standard si traspone, in tutta evidenza, nel presente provvedimento. la grande questione economico-tributaria. Dal punto di vista complessivo, questo schema di decreto potrebbe potenzialmente determinare un aumento assai significativo del prelievo fiscale a carico dei cittadini. Tali nuove imposte non fanno che tradire sotto il profilo strettamente normativo la legge madre sul federalismo fiscale: non era, infatti, prevista l'introduzione di alcuna nuova imposta. la garanzia della «determinazione periodica del limite massimo della pressione fiscale nonché del suo riparto tra i diversi livelli di governo», oltreché la salvaguardia «dell'obiettivo di non produrre aumenti della pressione fiscale complessiva anche nel corso della fase transitoria». L'aumento potenziale della pressione fiscale complessiva del presente decreto è dimostrata, in modo chiaro ed inequivocabile, anche dal non accoglimento, da parte del Governo e della maggioranza, della proposta emendativa n. 21, presentata dal nostro Gruppo parlamentare, proposta che mirava proprio alla sua invarianza tributaria. Per questo, Signor Ministro, siamo spiacenti di non poter votare a favore del federalismo municipale. Se perfino il presidente della Corte dei conti, Luigi Giampaolino, che non è certo vicino alle posizioni nostre e dell'opposizione, ha sottolineato il rischio, durante il suo discorso in apertura dell'anno giudiziario, che che l'impianto del federalismo possa produrre squilibri interni e dislocazione territoriale del gettito fiscale e incertezza sulla sua effettiva invarianza, ciò vorrà pur dire che le nostre osservazioni non sono infondate. Giampaolino ha ricordato, come già detto, che lo schema iniziale di decreto «prefigura il nuovo sistema di finanziamento delle amministrazioni comunali basato non più su trasferimenti erariali bensì, in via prioritaria, sui proventi della tassazione immobiliare fino ad ora solo in parte di competenza comunale» e la definizione del nuovo tributo, l'IMU, in sostituzione di una serie di prelievi diretti e indiretti che gravano sul reddito da immobili.

ma è stata posta, comunque, l'attenzione su alcune osservazioni critiche di carattere generale attinenti sostanzialmente alla coerenza del disegno con gli obiettivi ed i criteri della legge delega, alla reale fattibilità dei risultati attesi e alla sostenibilità delle soluzioni proposte». Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa o il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, stessi. Inoltre, questo decreto sblocca l'addizionale IRPEF già dal 2011, senza attendere l'entrata a regime della compartecipazione all'IRPEF del 2 per cento Nel frattempo, i Comuni possono istituire o aumentare l'addizionale fino allo 0,2 per cento e possono aumentare l'addizionale anche retroattivamente, a valere sul 2010.

Chi ci guadagnerà nell'immediato saranno i proprietari di immobili con i redditi più elevati e non è scontato che, nel lungo periodo, possa servire a incoraggiare l'emersione dei canoni irregolari o in nero.

all'imposta di soggiorno. Si tratta di una tassa odiosa, signor Ministro. Tale imposta, inizialmente prevista per i capoluoghi di provincia, è stata estesa a tutti i Comuni turistici e gli introiti dovrebbero essere destinati alla manutenzione e al recupero dei beni culturali e ambientali e ai servizi pubblici locali. Siamo nettamente contrari perché, oltre ad essere una tassa ulteriore che viene addossata ai cittadini, avrà un effetto deprimente sul turismo, in un momento in cui il Paese ha bisogno di crescita ed il comparto del turismo è uno di quelli che può dare un contributo importante alla ripresa dello sviluppo. Questo ulteriore balzello va contro uno dei principi fondamentali che avevano portato l'Italia dei Valori a votare a favore della legge delega sul federalismo fiscale: la responsabilizzazione degli amministratori. Pagheranno, infatti, la tassa coloro che non saranno mai chiamati a giudicare attraverso il voto gli amministratori che hanno utilizzato quei denari. La compartecipazione all'IVA è l'ultima modifica introdotta dal decreto. È prevista una compartecipazione all'IVA dei Comuni, ma la percentuale non è stata definita ed è rinviata ad un decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri. alla tassa di scopo, i Comuni potranno finanziare specifiche opere pubbliche richiedendo un contributo ai cittadini. Anche i piccoli Comuni, signor Ministro, denunciano il precario equilibrio in cui versano i loro bilanci,

*(PD)*. Signora Presidente, il decreto legislativo al nostro esame sul federalismo fiscale municipale viola i principi fondamentali stessi di un ben ordinato assetto federale sotto il profilo del fisco. Quel ben ordinato assetto federale dal punto di vista fiscale che abbiamo scritto in Costituzione con l'articolo 119 e che voi della maggioranza di centrodestra dovete aver giudicato condivisibile, anzi del tutto condivisibile. Infatti, nel corso di un'attività di riforma della Costituzione molto radicale a cui avete dato vita nel corso della legislatura tra il 2001 e il 2006, l'unico articolo che è sopravvissuto intatto a quel tipo di iniziativa riformatrice è proprio l'articolo 119: se avete modificato tutti gli altri e non avete cambiato questo, devo dedurre che vi piacesse, che avesse da parte vostra un giudizio positivo. Ebbene, la mia tesi è che che la soluzione da voi adottata sul federalismo municipale vìoli i princìpi fondamentali cui dovrebbe ispirarsi una buona iniziativa attuatrice dell'articolo 119 della Costituzione.

quale chi è titolare del potere di spendere è titolare del dovere di reperire nell'economia e nella società le risorse necessarie per effettuare quella spesa. Il regime vigente, fondato sui trasferimenti da parte dello Stato centrale al sistema delle autonomie (dal centro alla periferia) e sulla centralizzazione assoluta del prelievo fiscale, è

e per quanto, sappiamo bene, della spesa pubblica sono responsabili gli enti locali - non è responsabile direttamente del reperimento delle risorse per realizzare quella spesa. Ma il problema, signor Ministro, è che il decreto in esame è altrettanto in opposizione a questo principio, poiché si limita a chiamare i trasferimenti di un tempo, ossia quelli attualmente in vigore, "compartecipazioni": battezza i trasferimenti "compartecipazioni", ma non cambia la natura del sistema applicando il principio di responsabilità, non afferma, cioè, la responsabilità dei sindaci sul prelievo

il mondo occidentale, quale che sia l'assetto - federale o non federale - del sistema, se vi è autonomia impositiva e finanziaria dei Comuni, o di ciò che è assimilabile ai nostri Comuni, questa è fondata sul prelievo sugli immobili. Chiunque si sia occupato di tale materia sa che le cose stanno così: in tutto il mondo, ma in Italia no, nemmeno attuando il provvedimento sul federalismo, che pure questo principio richiama con grande nettezza. Perché no?

non condivido tale scelta, ma la comprendo. Ma perché, per tenere fede a questa scelta, ostinatamente vi rifiutate di applicare al decreto sul federalismo municipale la soluzione adottata in tutto il mondo? Il prelievo dell'imposta municipale inerisce a tutte le case, a tutti gli immobili che stanno in quel dato Comune: poi, naturalmente, se per scelta politica si vuole completamente esentare la prima casa da quel prelievo, si consentirà al cittadino, alla famiglia, di realizzare una detrazione pari al tributo pagato. Non cambia assolutamente niente sotto il profilo finanziario, ma si afferma il principio. posizioni parassitarie dei Comuni, cioè i tentativi di azzardo morale su questo versante, sarebbe facile combatterle con misure che vi abbiamo anche proposto, per cui quello che ha detto nella relazione su questo punto, mi consenta, signor Ministro, è completamente destituito di fondamento tecnico. Secondo elemento di violazione di principio fondamentale: questo decreto viola il principio, sacro per la democrazia parlamentare rappresentativa, secondo cui c'è un legame indissolubile tra tassazione e rappresentanza. «Nessuna tassazione senza rappresentanza» imposero, molti secoli orsono, coloro che diedero vita al primo dei Parlamenti che noi possiamo considerare antenati delle nostre democrazie parlamentari. Nessuna tassazione senza rappresentanza. Ora, questo decreto stabilisce che l'imposta comunale fondamentale verrà a considerare come propria fondamentale base imponibile le seconde case. Siamo in presenza di un evento storico, cioè del rovesciamento del principio fondamentale su cui si è fondata la democrazia parlamentare. Qui, secondo il Governo, applicando nientemeno che il federalismo fiscale, dobbiamo realizzare, credo unico Paese al mondo, il principio secondo cui c'è tassazione ma non c'è rappresentanza. tassazione ma non c'è rappresentanza. Infatti, chi vota per il sindaco non pagherà le tasse definite dal sindaco, perché è abitante di quel Comune e ha lì la prima casa e non la seconda,

Noi abbiamo un sistema fiscale (qui stiamo parlando di fisco) decisamente sperequato: la pressione è troppo forte sul lavoro, troppo forte sul reddito d'impresa e troppo debole su altre basi imponibili. Tutti lo diciamo. E poi, guardiamo questo decreto, che sblocca l'addizionale IRPEF per i Comuni. Certo, i Comuni hanno richiesto questo sblocco, e io li capisco: dal punto di vista sindacale è chiaro che il mio amico Chiamparino e tutti

Questa addizionale IRPEF è un aumento di pressione fiscale a cui i Comuni saranno costretti sul lavoro: quindi, «più sul lavoro e meno sulla rendita», perché nella proposta dell'IMU c'è un'evidente patrimonializzazione dell'IRPEF pagata sugli immobili non locati. Il decreto, per di più, prevede una forte agevolazione, del 50 per cento dell'aliquota, per gli immobili locati che pagheranno la cedolare, e questo è anche giusto,

risultato è che voi spostate prelievo dalla rendita verso il lavoro e l'impresa, il contrario di quello che affermate sotto il profilo dei principi generali.

è una richiesta che avanziamo da anni. Ma essa non farà emergere base imponibile se non si sposa - come nel decreto non si sposa, per vostro pervicace rifiuto

nel famoso Nord, al bar lo sanno tutti che va così. C'è convergenza degli interessi? Allora funziona. Non c'è convergenza di interessi? Non funzionerà. Risultato: questa

signor Ministro: per il merito di questo provvedimento, non perché essere contro serve per vedere se riusciamo a far cadere Berlusconi. Noi vogliamo far cadere Berlusconi, ma questo è un altro paio di maniche: abbiamo dimostrato che abbiamo saputo tenere fuori il tema del federalismo fiscale. Siccome l'articolo 119 è un nostro articolo, almeno tanto quanto vostro, anzi di più, quindi abbiamo fatto uno sforzo politico serio per tenere fuori l'attuazione dell'articolo 119 dal conflitto maggioranza-opposizione, oggi asperrimo, che ha per oggetto la caduta del Governo. Siete voi che ci avete imposto, con soluzioni di merito letteralmente assurde, un voto contrario, che non a caso sulla legge non abbiamo espresso, perché la legge invece è stata oggetto di un confronto positivo che ha dimostrato che siete voi che state strumentalizzando il tema del federalismo fiscale per fare la respirazione bocca a bocca ad un Governo che è un organismo morente. Noi diamo una valutazione sul merito e, sulla base di questo giudizio di merito, esprimiamo il nostro voto contrario.

ma il ritardo della mancata riforma dello Stato centrale ha prodotto una seria inefficienza dell'apparato pubblico a tutti i livelli, a danno dei cittadini, delle famiglie e delle imprese, sulle cui spalle sono ricaduti poi i costi relativi. Se non si procede con questa importante riforma in maniera organica, uniforme e bilanciata, con un debito pubblico come il nostro e con una crescita economica che, per vari motivi, è spenta e comunque è bloccata, potremmo veramente rischiare di finire nel baratro. È certo che l'elezione diretta dei sindaci e dei governatori e la riforma del Titolo V della Costituzione del 2001 hanno conferito agli amministratori locali maggiori poteri, e questi però, con le casse sempre più vuote, hanno di fatto scaricato sui cittadini i costi del Governo centrale, con il risultato di una maggiore pressione fiscale complessiva. È quindi evidente la necessità di agevolare le potenzialità delle piccole e medie imprese, che sono la vera spina dorsale dei nostri territori. In Inghilterra, il primo ministro Cameron parla di «grande società», progetto politico che concepisce la comunità come protagonista della modernizzazione, sulla base di due linee guida: la libera iniziativa e la solidarietà attraverso la decentralizzazione. In Italia, in che modo deve avvenire questa modernizzazione? In che modo possiamo uscire dalla crisi economica più forti di prima? Certo non con questa soluzione di federalismo. L'Unione di Centro conferma, coerentemente, la propria opinione contraria su questa impostazione di federalismo fiscale. Come può essere credibile, infatti, un federalismo nel quale non si sa "chi fa che cosa" e nel quale non sono definiti i livelli essenziali delle prestazioni con cui lo Stato deve garantire a tutti a tutti i cittadini le risorse possibili? Come può essere credibile un federalismo in cui le funzioni fondamentali degli enti locali sono definite soltanto in maniera forfetaria? Questo è un federalismo senza numeri, del quale non si conosce nulla, e soprattutto questo è quello che ci preoccupa. E, a proposito di imposte, crediamo che queste debbano riguardare solo il cittadino residente, rispettando così il principio cardine che sancisce il legame indissolubile tra amministratore e amministrato, rafforzandone di conseguenza la responsabilità. Per quanto riguarda il *modus operandi* di questa riforma, sarebbe stato innanzitutto indispensabile e opportuno, prima di procedere all'attuazione del federalismo fiscale, modellare il sistema istituzionale rendendolo veramente federalista; stabilire le competenze dei vari livelli di governo in modo da chiarire di chi sono le responsabilità e su chi ricadono gli oneri. Solo allora sarebbe stato opportuno aprire il dibattito sul federalismo fiscale, che non può che essere considerato solo una parte, ma quella conclusiva, di una più ampia ed organica riforma istituzionale. In questo provvediménto ci sono molte cose che non vanno: la mancanza dei dati relativi al gettito derivante dalla fiscalità immobiliare; la compartecipazione all'IVA attribuita ai Comuni; la cedolare secca, che premia i redditi alti a scapito di tutti quelli bassi; mancata previsione di agevolazioni per le famiglie con figli; l'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive, che graverà pesantemente sul settore del turismo e non rappresenta di certo uno stimolo per il settore stesso; l'imposta di scopo, che farà gravare sui cittadini il finanziamento delle opere pubbliche realizzate dai Comuni, e tutte le altre nuove forme di imposizione fiscale sostitutive, che finiranno per aumentare la pressione fiscale sulle famiglie e sulle imprese. Signor Ministro, noi abbiamo un'idea diversa del federalismo fiscale: competenze e funzioni chiare e nette dello Stato, delle Regioni e delle autonomie; un ruolo insostituibile dello Stato nella perequazione e nelle politiche di sviluppo economico e di coesione sociale. Per questo, noi dell'UDC abbiamo deciso di assumere una posizione contraria a questo federalismo, che consideriamo pericoloso e iniquo, almeno fino a quando non saranno garantite a tutte le Regioni del nostro Paese le stesse opportunità e le stesse occasioni di sviluppo.

senatore Vaccari.

ci conosciamo, e quindi immagino anche quello che poteva comunicarci. Comunque, signora Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi,

di completamento legislativo che ha visto prima la legge n. 42 del 2009, dopo solo un anno di insediamento da parte di questo Governo e di questa maggioranza, e poi tutti i decreti delegati collegati che man mano si stanno sviluppando. come mai da parte del PD vi sia questa posizione di fermarsi, di essere un partito conservatore, di non voler cambiare nulla, di votare sempre no, o formalmente no, anche nei casi in cui molte delle proposte formulate sono state anche accolte, inserite nei testi sia durante della legge delega principale di indirizzo, sia durante l'esame dei vari decreti attuativi. A tale proposito devo dare atto al ministro Calderoli di aver sempre tenuto una posizione molto aperta, molto disponibile con tutto l'arco costituzionale della Camera e del Senato proprio perché questa è l'esigenza e la richiesta che ci viene da tutto il Paese, un Paese che è diviso e disunito e che può trovare e trova solo tramite il federalismo - come bene ha detto il Ministro nella sua relazione - la sua unione, la sua possibilità di ricollegarsi. Ecco che quindi noi diciamo di andare avanti in questa direzione. Quando un popolo è in cammino, questo popolo può piegare la storia. Gli esempi sono eclatanti anche sullo scenario mediterraneo, purtroppo lì con violenze e con conflitti. Certamente guardiamo con preoccupazione a quanto sta avvenendo. Il movimento che stiamo facendo noi è di tipo democratico, è voluto dalla gente e va verso questo forte cambiamento. Tra l'altro, come amministratore, ho l'onore e l'orgoglio di essere sindaco di una città, Feltre, e non vedo l'ora di poter applicare subito queste possibilità di autonomia, di passare da questa finanza derivata a una finanza appunto di autonomia, potermi mettere in gioco anche nei confronti dei miei cittadini, di capire quali sono gli strumenti migliori, come modularli e passare alle varie manovre e alle varie leve che ha l'amministrazione locale

Solo questo può far pensare a quali possono essere le emersioni del nero esistente in alcune parti del Paese, il riequilibrio, che tutti desiderano, sul pagamento delle tasse e sulla partecipazione

Signor Presidente, signor Ministro, signori membri del Governo, onorevoli colleghi, oggi è grande la soddisfazione di poter intervenire e confrontarci su questo tema importante del federalismo municipale, che non sta a cuore soltanto alla Lega Nord, alla maggioranza e a quelle forze politiche responsabili che siedono in Parlamento, ma rappresenta assolutamente un altro paso fondamentale per il rinnovamento di questo Paese.

il federalismo fiscale, attraverso gli otto decreti legislativi, all'insegna dell'autonomia e della responsabilità. I protagonisti diventano i Comuni, le Province, le Regioni.

Si sta lavorando sul ruolo di un ente intermedio, che ha un senso nel momento stesso in cui diventa un riferimento per il territorio. Quindi l'abolizione di tutte le Province in genere? Assolutamente no.

una precisazione che ritenevo importante fare. Voglio riferirmi a quanto detto, nella sua relazione molto dettagliata, dal ministro Calderoli. Oggi, con questo decreto, passiamo dalla finanza derivata a quella autonoma, sostituendo oltre oltre 11 miliardi di trasferimenti statali annui, assegnati, come dicevo prima, in base al criterio, assolutamente irrazionale, della spesa storica. Tutto questo viene sostituito con tributi propri e compartecipazioni.

non è così. Dal 2014, come ha detto il Ministro, alcuni tributi statali sono assorbiti nelle imposte municipali propria e secondaria, senza nessun aggravio per il contribuente. Il decreto sul fisco comunale riduce

municipale. Sono certo che le votazioni di domani in quest'Aula evidenzieranno la condivisione che esiste sul federalismo, che deve dare delle risposte concrete al territorio, ai Comuni, ma soprattutto ai nostri cittadini.

collega Morando, chiarisce in modo esplicito quali sono i confini all'interno dei quali deve operare il federalismo perché possa funzionare. Uno strumento fondamentale, se fatto bene, per combattere gli sprechi, attraverso la responsabilizzazione degli amministratori locali, e per combattere l'evasione, proprio attraverso il fatto che si avvicina il luogo in cui viene eseguito il Nella realtà questo non c'è. Lei, Ministro, ha parlato del famoso «pago, vedo, voto», ma non capisco dove sia, non lo trovo, nel senso che le tasse continueranno ad arrivare a Roma, da dove ritorneranno poi sul territorio, mediate dal fondo perequativo, che diventa così una "centrifuga", una "lavatrice", che alla fine impedisce di avere di fatto la tracciabilità delle risorse prodotte da quel territorio. Questo è un dato non indifferente.

Ci sono contribuenti che pagano oltre il 50 per cento del loro reddito: punti pagheranno ancora di più, mentre gli evasori non pagheranno nulla. Questo è il problema di questo federalismo.

ai possessori di immobili (di seconde case), ai possessori di attività o ai percettori di reddito IRPEF, e agli altri nulla, secondo voi, un condominio così organizzato

qua siamo «commissariati in casa nostra». I Municipi non sono più quelli di una volta: c'era più autonomia dieci anni fa. Questa è la realtà, e ve lo dice un ex sindaco: nel 2003 c'era più autonomia che nel 2011. Al riguardo, vi sfido con delle proposte concrete, che mettono al centro queste questioni: innanzitutto, l'eliminazione dell'addizionale IRPEF. Questa è una proposta seria: eliminare l'addizionale IRPEF, che significa abbassare la pressione fiscale per i contribuenti onesti.

Sono come i soldi presi alla lotteria: si rischia di spenderli male. Altra cosa sono le risorse che il sindaco, con la sua faccia, che è quella del Consiglio comunale e della maggioranza, deve chiedere ai suoi cittadini per dare dei servizi, e per darli nel miglior modo possibile.

Questo è il problema. Perché non volete i nostri voti per fare un federalismo fatto bene e preferite fare un federalismo clientelare, che anche nel milleproroghe è andato a dare vantaggi clientelari alle Regioni «speciali», «speciali», che da questo decreto non vengono assolutamente toccate? Questo è federalismo clientelare, e noi non abbiamo più la possibilità di fare clientele in un Paese che, come giustamente ricordava prima il collega Massimo Garavaglia, ha un debito pubblico di 1.860 miliardi di euro.

Questo è il federalismo che volevamo? Questo è il federalismo che abbiamo promesso? No: né voi della Lega, né voi del Popolo della Libertà, né noi del Partito Democratico. Non abbiamo promesso questo. Abbiamo promesso di portare più equità e giustizia nella distribuzione delle risorse;

che mirano proprio a realizzare tale obiettivo. C'è una proposta di risoluzione a mia prima firma che si pone come obiettivo quello di responsabilizzare di più gli enti locali e gli amministratori locali, dando loro maggiore autonomia finanziaria.

attenzione questo decreto legislativo, come i precedenti, e di aver cercato fino in fondo di trovare le possibili mediazioni in una materia molto delicata e molto condizionata da

Ho avuto la sensazione che il giudizio delle opposizioni sia stato negativo soprattutto perché condizionato da fattori politici, nella convinzione che il negare il parere favorevole a questo provvedimento significasse la caduta del Governo

purtroppo tra pochi intimi ad esprimere un parere su questo decreto legislativo, come richiestoci dal Presidente della Repubblica. Credo che questo decreto legislativo sia quello che è possibile fare in questo momento. È certo che si poteva fare di molto meglio, ma ci sono due limiti che condizionano fortemente l'impostazione di questo decreto. Da un lato, nessuna forza politica, salvo in qualche modo il senatore Baldassarri, ha avuto il coraggio di dire francamente che bisognava nuovamente reintrodurre in questo decreto legislativo, anche in modo surrettizio o in modo nuovo. L'ICI Tutti, per ragioni popolari, politiche e di consenso, hanno sostenuto (e sfido qualcuno a dimostrare il contrario) che non si doveva introdurre alcuna tassazione sulla prima casa. Questo obiettivamente è stato uno dei limiti strutturali del provvedimento. È chiaro infatti che se si vuole impostare un federalismo municipale adeguato bisognerebbe tener conto di tutte le case, comprese le prime,

è poi completata con l'intervento del Governo Berlusconi, ha fatto sì che oggi questa questione sia un tabù. Come secondo

Regioni. Infatti, sono sempre più convinto che dovrebbero essere le Regioni a detenere la regia della distribuzione delle risorse, delle compartecipazioni e dei fondi perequativi, e che non debba essere lo Stato, riesco ad immaginare come si riuscirà a ripartire il fondo perequativo di riequilibrio tra tutti i Comuni d'Italia, dal Nord al Sud: è una cosa complicatissima, mentre, se tutto venisse gestito a livello regionale, sarebbe più semplice. Ne ho avuto esperienza diretta, essendo stato lungamente amministratore regionale del Friuli-Venezia Giulia: siamo riusciti,

pertanto, questo decreto va visto in questa logica, con i vincoli politici sulla prima casa e i vincoli costituzionali. In secondo luogo, questo è un primo passo. Qui si chiede sostanzialmente di non fare niente per fare le cose più perfette, ma andando avanti sulla linea del ricercare la perfezione non si fa niente. Sono convinto che sia meglio partire poi, dalla sperimentazione che si farà nelle varie aree del Paese, si arriverà a trovare le soluzioni migliori, mi auguro anche in un quadro di cambiamento della Costituzione in modo da consentire veramente di ristrutturare il Paese su base federale con un ruolo centrale delle Regioni nel rapporto con gli enti

la situazione potrebbe diventare devastante. Quanto regge ancora nel nostro Paese la possibilità di trasferire dal Centro-Nord, dalle aree economicamente più importanti e competitive del Paese,

una situazione economica che ogni anno consentiva di aumentare il prodotto interno lordo. Oggi, con i vincoli di debito e con la caduta della crescita economica, queste ulteriori possibilità di trasferimento di

a favore delle popolazioni che le producono, e non certamente continuare in una situazione che ci ha portato a finanziare tante inefficienze che sono sotto gli occhi di tutti. di tutti. Qui si è molto puntato sul recupero del ruolo da parte delle amministrazioni comunali in materia di evasione fiscale. Nel 1975 ero un giovanissimo sindaco. Erano gli anni in cui si è applicato il decreto Stammati. si applicavano perché non era più possibile gestire a livello locale l'imposta di famiglia. Venivano fuori delle guerre nei Comuni perché le Giunte e i Consigli comunali applicavano

fiscale ci sarà solo sulla questione della cedolare secca, anche perché oggi gli strumenti informatici a disposizione quarant'anni dopo, rispetto a quando si sono applicati i decreti Stammati sono del tutto diversi. Oggi

tenendo conto che questo è un provvedimento certamente importante, una sperimentazione, che potrà essere migliorato in futuro. Bisogna però tenere conto di una cosa. Quest'anno ricorre il 150º anniversario dell'Unità d'Italia,

La risposta a questa Unità d'Italia che non è mai nata veramente è costruire un sistema federale nuovo. Ho la preoccupazione che, se ci attarderemo ancora nel processo riformatore,

ma soprattutto perché a un certo punto i cittadini del Nord produttivo, della Slovenia e della Croazia, non ritenevano più di dover mantenere il potere centralizzato serbo. È scattata così la rottura e la deflagrazione in quel Paese. Anche noi, in una situazione economica, finanziaria e istituzionale molto delicata come quella che stiamo

il ministro Calderoli - noi dell'Italia dei Valori siamo ancora più convinti che con questo decreto ci viene proposto un ulteriore passo indietro di un federalismo alla rovescia, un federalismo che ci sta consegnando, anche in questa occasione,

Dicevo che ci ha regalato, signor Ministro, anche con questo decreto, una nuova scatola vuota dove l'indeterminatezza dei contenuti e delle cifre dell'impatto finanziario ha, di fatto, prodotto una regressione rispetto alle finalità della stessa legge delega nella quale, come lei sa, noi dell'Italia dei Valori abbiamo votato favorevolmente. Il primo problema è l'ambiguità del decreto: dice poco su quello che avverrà da qui al 2014, e poco più di nulla su quello che succederà dal 2014 in poi. Nella formulazione dei decreti precedenti, che sono, come lei sa, signor Ministro, cosa ben diversa dalla loro attuazione, da un lato viene rinviata la definizione dei fabbisogni *standard* agli studi successivi della SOSE e dall'altro - cosa per noi abbastanza grave - si opera nella totale ignoranza del fatto che i costi standard sono il vero parametro di riferimento per la determinazione delle risorse, per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni Il decreto che discutiamo oggi aggrava ulteriormente questa impostazione, legando le risorse dei Comuni al gettito di un insieme di imposte. In sostanza, si rivela per quello che non doveva assolutamente essere: un riaggiustamento di un sistema di decentramento fiscale, che altro non è che un modesto riassetto fiscale.

si crea una compartecipazione sulla tassazione erariale dei trasferimenti immobiliari, si introduce, con la cedolare secca, un'imposta sostitutiva dell'IRPEF sugli affitti. Di fatto questa presunta riforma si esaurisce in uno spostamento del carico fiscale - diciamolo sino in fondo - dai proprietari di case, quelle date in locazione, alle imprese e ai lavoratori autonomi. E l'unica cosa veramente importante per ricreare un rapporto stretto di responsabilità tra amministratori e cittadini (come ha ricordato il Ministro nella sua relazione), è il fatto di riportare a tassazione la proprietà della prima casa, non si è avuto il coraggio di affrontarla. Allora, restano del tutto irrisolti alcuni nodi di fondo. Ne cito due: la limitata autonomia riconosciuta ai Comuni, con la riduzione di fatto (e lo vedremo) delle risorse complessive; l'assenza di una risorse complessive; l'assenza di una regolamentazione certa e coordinata del sistema perequativo dei Comuni, perché restano del tutto indeterminati gli effetti redistributivi del nuovo finanziamento municipale, non solo tra tipologie di Comuni (i cosiddetti Comuni virtuosi e quelli che, a giudizio della Lega Nord, non lo sono), ma tra territori diversi e quindi ancora di più tra Nord e Sud. Andiamo per ordine ed entriamo nel merito di alcune questioni che, a nostro giudizio, hanno una ricaduta nulla, se non addirittura negativa, sulle politiche concrete. Gli spazi di autonomia tributaria dei Comuni rimangono quasi nulli (intendiamoci su tale aspetto prima di andare avanti), perché fino al 2013 non avranno alcuna autonomia decisionale sulle aliquote dei tributi loro assegnati

molti Comuni saranno costretti ad aumentare le addizionali IRPEF per recuperare almeno parte delle minori entrate. Questa non è una denuncia di parte.

scriva: «Nello specifico della problematica del coinvolgimento delle autonomie territoriali nella programmazione economico-finanziaria, si sottolinea una certa vaghezza della formulazione normativa

Dal 2014 in poi, il principale tributo proprio dei Comuni verrà pagato prevalentemente da soggetti non residenti, accentuando ancora di più la contraddizione aperta dall'abolizione dell'ICI sulla prima casa.

e più tasse per i redditi da lavoro e da pensione per effetto dello sblocco parziale delle addizionali IRPEF, mentre sarà notevolmente ridotta l'imposizione sui proprietari di immobili locati grazie all'introduzione della cedolare secca sugli affitti.

almeno due problemi. Il primo riguarda la perdita di gettito derivante dallo sconto fiscale riconosciuto ai contribuenti e che difficilmente sarà compensata, in termini di neutralità finanziaria, dall'ipotesi

Il secondo problema della cedolare secca è rappresentato dal fatto che è quanto meno discutibile che il Governo voglia destinare risorse così rilevanti alla riduzione dell'imposizione fiscale sui proprietari di immobili, con benefici,

L'altra grande questione che abbiamo sollevato nel nostro lavoro in Commissione riguarda le modalità di alimentazione e di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio,

avverrà in base ai fabbisogni *standard* o alla capacità fiscale degli enti. Cosa succede al fondo di riequilibrio e alla perequazione tra i Comuni? Non lo sappiamo perché il decreto non lo dice. Come si fa poi a calcolare esattamente quanta parte del gettito IMU di un Comune deve tornare al fondo perequativo? Chi e in che modo lo decide? Non lo sappiamo perché il decreto questo non lo dice. E se poi i tributi confluiti nell'IMU finiscono interamente nelle casse comunali, i Comuni che presentano ricchezza immobiliare nelle seconde case, avranno oggettivamente (questo è un dato di fatto) un sistema che li avvantaggerà rispetto agli altri territori.

Signor Ministro, se mi consente, per la stima e la simpatia che le portiamo, le consigliamo di leggere un buon testo, un testo del professor Gianfranco Viesti, il quale usa una espressione che per noi vale come raccomandazione che rivolgiamo al Governo.

- «ma domani negli effetti virtuosi che deve produrre». Noi di questi effetti non vediamo nessuna traccia. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, signor Sottosegretario, in ogni buona discussione accademica (tale mi pare questa, anche per l'effetto che poi avrà domani sul voto), c'è sempre qualcuno che ha la testa più dura degli altri e resta sempre un passo indietro. Adesso tocca a me: abbiate pazienza, perché sono rimasto un passo indietro. Federalismo fiscale: è vero che l'ottimo è nemico del bene, ma certo, a me pare, tentare di mettere insieme due riforme mancate per produrne una è qualcosa di più di un ottimo da ricercare. Perché il federalismo è una riforma mancata? Perché se ne parla in termini di federalismo fiscale quando mi sarei aspettato

federale dello Stato. Ancorché si possa discutere sul processo storico (gli Stati federali nascono per mettere insieme pezzi che vogliono stare insieme e non stavano insieme per la nostra Repubblica mi sembrerebbe difficile immaginare quel percorso storico), mettiamo che occorra disegnare lo Stato veramente più moderno, più efficiente, più efficace, come ho sentito dire, più snello. Allora mi sarei aspettato una impostazione federalista avrei incominciato a togliere degli elementi che rendono lo Stato così pesante. Quanti livelli decisionali e di spesa ci devono essere in uno Stato?

un gesto realmente coraggioso, ancorché coerente con cose che erano state dette da questo Governo in campagna elettorale, e condivise anche da tantissimi altri, anche dell'opposizione. A proposito di allargamento della maggioranza, qualcuno qualcuno mi spiega perché non si riesce a portare avanti quel disegno così interessante dell'abolizione delle Province? Signor Ministro, lei ha Signor Ministro, lei ha scritto autorevolmente che questo si può fare nell'invarianza della Costituzione: ha scritto un articolo, secondo me bellissimo, in cui spiegava come si poteva tranquillamente lasciare le Province senza il peso della politica. Perché non si può fare? Eppure, quanti siamo? Tutti a dire che vorremmo questo. Potreste verificare in effetti se la maggioranza in questo ambito è allargata. Ma non succede niente sotto questo profilo, anzi, mi pare addirittura vi sia qualche marcetta indietro! Mi sembra che lo Stato non si snellisca, non vada verso lo Stato federalista, dei pezzi di Stato che si uniscono insieme: che senso avrà mantenere ancora le Regioni a statuto speciale? Perché non si disegna quello? «Fiscale»: ma non avrebbe avuto senso incominciare a ragionare finalmente di qualcosa di cui tanti, tutti parliamo da tempo, cioè della riforma del fisco in questo Paese? Perché anche questa è una riforma che manca. si arrabatta su temi fiscali in atto, quando ci sarebbe bisogno di ridisegnare il fisco sul piano delle famiglie e delle imprese. Mi

che questo abbia una sua logica: mi sembrerebbero musica e parole più comprensibili, più semplici, più orecchiabili, più spiegabili.

Però, bisognerebbe riuscire anche a spiegare perché alcune cose che si è detto si sarebbero fatte non si fanno, eppure erano in quel segno: perché adesso se ne fa un'altra? Non so, a me pare che, se l'ottimo è nemico del bene, forse ci sono parole e musica, a proposito di canzoni (siamo ancora in clima festivaliero), che sarebbero suonate meglio. Io avrei ricominciato da parole scritte nella Costituzione. La nostra Costituzione usa poche volte un verbo a mio avviso di straordinaria importanza: è il verbo riconoscere. Vuol dire che vede cose che ci sono già, prima che siano scritte. Lo usa per i diritti e lo usa poi per le autonomie: «La Repubblica (...) riconosce e promuove le autonomie locali». Io avrei cominciato da lì.

di più. Tutti avremmo dovuto partecipare con un sano trasversalismo, come è stato ricordato poc'anzi, all'elaborazione di questa riforma che riguarda tutti. Fintanto che in questo Paese non scopriremo che la riforma non riguarda solo la Lega, il PdL o altri partiti, ma riguarda tutti, credo che non faremo alcun passo avanti.

perché non sto a ripetere che il federalismo è altra cosa, ma dico quello che ha detto l'altro ieri il presidente della Corte costituzionale italiana, quale ha detto che il federalismo è una bestemmia nell'attuale assetto costituzionale. Si tratta di uno Stato delle autonomie, come ricordava il senatore Gustavino. Le ricordo anche che voi avete avuto dei contrasti forti con il professor Miglio

ti do questo e tu mi dai quello. No! Su queste cose il mercato non deve avvenire. Facciamolo su altre, ma mai sulle riforme, e in particolare su questa grande riforma dello Stato che stiamo portando avanti. accreditare in alcune parti della popolazione italiana che il federalismo oggi - e non lo è, e poi lo vedremo - potrebbe trasformarsi esclusivamente in un egoismo territoriale. Ecco perché, signor Ministro,

è diventata una baraonda: chi tira la coperta a destra e chi a sinistra. Perché? Perché non vi sono regole certe. Il federalismo, quando ci sono regole, protegge soprattutto le popolazioni e le comunità più Mi dispiace. Anche l'*iter* in Commissione, così frettoloso, credo che sia stato un errore. Andava meditato e necessitava più coinvolgimento da parte del Parlamento. Il fatto che sia tornato in Parlamento per caso credo che sia l'occasione che ci viene data per fare alcune riflessioni aggiuntive sul federalismo.

È stato ricordato che sono stati tagliati oltre 2.100 miliardi. Credo che questa riforma cada in un momento di grande Oggi riconfermiamo che crediamo ad uno Stato delle autonomie, alla responsabilità degli amministratori, però vogliamo portare avanti anche il federalismo, o l'autonomia, istituzionale:

Io credo che sia importante partire, per poi chiudere, dall'attuale situazione finanziaria dei Comuni. È vero: non tutti forse sanno che, sotto il fascismo, i Comuni avevano più potere fiscale di oggi. oggi. Avevano entrate autonome molto, ma molto più cospicue di quelle di oggi. Man mano, la legislazione italiana negli anni è venuta a dare meno potere e meno autonomia finanziaria e fiscale ai Comuni.

al centro). Partendo da questo fatto, dire no alla spesa storica è un fatto positivo.

Uno Stato, sia pur autonomo, deve portare avanti una perequazione giusta che penalizzi, certamente, i cattivi amministratori. Ecco perché la vera sfida, che non è affrontata ‑ e me ne dispiace ‑ in questo decreto, è la sfida della perequazione. Addirittura, essa

Uno Stato unitario deve tener conto di una solidarietà fondamentale, che deve venir fuori, sì, sulla base della responsabilità degli amministratori, che devono porre fine agli sprechi (e lo ammettiamo, ce ne sono stati tanti, ma non solo nel Sud, credo): ma non si reagisce

non penalizzando, non a danno delle popolazioni povere. Riequilibriamo, invece, la spesa in base ai livelli essenziali delle prestazioni. Perché noi dobbiamo sapere quali sono i livelli essenziali delle prestazioni,

innanzituuto di dire che tutto il Gruppo della Lega Nord è orgoglioso di avere avuto oggi presenti in Aula tutti i rappresentanti di Governo della Lega Nord e, *in primis*, il nostro segretario federale, il ministro Umberto Bossi. Naturalmente siamo anche in un periodo abbastanza complesso e difficile, viste le crisi che in questi giorni si stanno manifestando con le rivoluzioni in atto. Sono trascorse appena tre settimane dal giorno in cui il Presidente della Repubblica giudicò irricevibile il decreto legislativo sul federalismo fiscale oggettivamente riscontrando quella forzatura procedurale frutto dell'*impasse* in cui venne a trovarsi la cosiddetta bicameralina. Allora, l'opposizione salutò quella sosta obbligata come la pietra tombale del Governo e del cambiamento: euforia svanita però rapidamente, visto che oggi siamo qui con un Esecutivo ben ben lungi dalla resa, una maggioranza rafforzata ed il federalismo che procede. Credo che occorra prendere atto di questa realtà, perché trincerarsi dietro aspettative velleitarie conduce ad atteggiamenti talmente pregiudiziali da vanificare quella disponibilità al confronto responsabile altrimenti auspicabile, trattandosi di una riforma della portata e rilevanza dell'attuale. Nessuno può imputare alla Lega Nord alcuna preclusione al dialogo, che abbiamo ostinatamente cercato e, a volte, persino inseguito. Nessuno - e lo dimostra anche il ruolo che l'ANCI ha avuto nella riformulazione del testo - può accusarci di insensibilità di fronte alle richieste di correzioni, più o meno condivise: un'apertura motivata dalla consapevolezza che una riforma di questa rilevanza riguardi tutti e che ciascuno debba sentirsene partecipe. Vorrei che risultasse chiara l'importanza del passaggio che stiamo affrontando, sancendo la nascita del federalismo municipale. Non si tratta, colleghi senatori, della semplice fase di un *iter* meramente preliminare agli altri quattro decreti, tra cui quello sul fisco regionale e provinciale. Con il federalismo comunale, infatti, ci troviamo alle sorgenti della rivoluzione federalista, alle fondamenta su cui poggia l'intero edificio. Non si compia l'errore di sottovalutare la centralità del momento.

Mi riferisco alla lapidaria sentenza del presidente della Corte costituzionale Ugo De Siervo, che ha addirittura definito «una bestemmia» il federalismo comunale, A suo avviso quello di cui ora stiamo trattando non sarebbe federalismo: secondo il Presidente della Consulta, «Dire federalismo municipale è una bestemmia: è come dire che un pesce è un cavallo, sono due cose che non stanno insieme».

Ebbene, l'affermazione del professor De Siervo ci aiuta a riconoscere quanto accade in questi giorni in quest'Aula, cioè che lo Stato italiano adempie nel 150° anniversario della sua unità al mandato morale ricevuto dagli artefici risorgimentali e mai ottemperato per un secolo e mezzo: l'unificazione federale di quegli Stati pre-unitari che, come dice De Siervo, godevano di piena sovranità, ma che furono annessi dal Regno centralista, *manu militari*, con l'avallo di ben dubbi *referendum.* L'unificazione federale, o perfino confederale, è quanto ci chiedevano i Cattaneo, i Rosmini, i Gioberti, i Ferrari. Oggi, tale processo parte propriamente dai Comuni, e non per intento blasfemo, ma semplicemente perché nella storia e nella cultura del nostro Paese il Comune è l'ente locale fondamentale. Sono i principi di autonomia e di indipendenza propri dell'età comunale che informano l'articolo 114 della Costituzione, là dove si sancisce che la Repubblica è costituita *in primis* dai Comuni, per aggiungervi successivamente «dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato». Precisamente dalla Costituzione italiana si evince che nel nostro Paese non può esservi il federalismo senza federalismo municipale; com'è assodato che, in difetto di una rivoluzione della finanza locale, qualsiasi rinnovamento istituzionale, ma anche morale, non produrrebbe esito alcuno. Concludo, signor Presidente, dicendo che il cambiamento procede e viene sancito dal federalismo municipale che sostituisce alla finanza derivata quella autonoma voltando pagina rispetto al malcostume dei trasferimenti statali assegnati in base al criterio della spesa storica. Non più cioè l'assuefazione ad una finanza locale drogata dai capitali a perdere piovuti dal Nord, ma una spesa pubblica in rapporto a valutazioni di efficienza e reperimento delle risorse anche da tributi propri e compartecipazioni. In definitiva, colleghi senatori, la responsabilità di chi amministra sul territorio, il rispetto della dignità di tutti i cittadini, del Nord e del Sud,

Signor Presidente, mi auguro che la discussione di oggi possa contribuire, se non altro, a smascherare la falsa rappresentazione che un'insistente, disinvolta ed abile propaganda della Lega ad accreditare (poc'anzi il ministro Calderoli, ma ne abbiamo avuto la plastica dimostrazione anche oggi perché i banchi del Governo sono occupati soltanto da rappresentanti della Lega e non abbiamo avuto il piacere di sentire interventi del resto della maggioranza,

cosa fatta, dando per sicuri, scontati ed acquisiti i risultati di portata storica per il contenimento della spesa, l'aumento dell'efficienza della pubblica amministrazione, il contrasto all'evasione, la riduzione della pressione fiscale. Tutte cose possibili, certo, ed anche contenute nell'impianto di principio e nella strumentazione attuativa prevista dalla legge n. 42, se però questa legge fosse stata attuata in modo coerente, rispettandone i presupposti, e non invece interpretata riduttivamente con dilazioni, omissioni e trascurandone aspetti fondamentali, come il caso del decreto di cui discutiamo è testimonianza. però sicuro che, se non altro, la nostra discussione servirà - almeno per me - a fornire una smentita netta su quello che considero un

che con riferimento alla qualità delle posizioni alternative e delle proposte avanzate al riguardo dal Partito Democratico e da tutte le opposizioni. Invito il ministro Calderoli a stare attento, perché deve esserci qualche zelante estensore delle osservazioni del Governo che hanno accompagnato il testo come presentato qui in Senato, anche se poi ho notato che lo stesso Ministro ha ripercorso più o meno la stessa traccia nella sua illustrazione di oggi.

Simone Simonini, artefice di documenti discutibili e di reinterpretazioni molto spesso fallaci che determinano effetti ed esiti poco positivi. È infatti strano aver tentato di ricostruire la discussione ed il voto dichiarato in Commissione bicamerale

Le cose infatti non stanno in questi termini. Lei sa benissimo che, per come era costruito il meccanismo tecnico, noi non potevamo fare altro che recuperare una parte dell'evoluzione del percorso della discussione, recependo parti del contenuto del parere di

Non ho difficoltà a riconoscere che lei, signor Ministro, si è sforzato di coinvolgere e di confrontarsi: ha avuto anche un atteggiamento dialogante. Però, sul merito non ci siamo intesi, e abbia la cortesia di riconoscere che noi non abbiamo presentato semplicemente delle proposte estemporanee, ma piuttosto delle proposte alternative di qualità. glielo dimostro ripercorrendo schematicamente per punti quelli che per noi sono elementi che inficiano l'impianto di questo provvedimento.

tutto è affidato a un fondo di riequilibrio per il quale - però - non ci sono criteri che garantiscono le modalità di riparto: è tutto rimesso alla genericità delle intese. Avete addirittura previsto alcuni criteri

Soprattutto, c'è un punto interrogativo inquietante sul 2013, l'anno che precede l'inizio della fase a regime. Ai Comuni avete già scippato i soldi che il decreto-legge n. 78 del 2010 ha tagliato e che avrebbero dovuto essere ripristinati.

caso la misura è valida. Tuttavia, il modo con cui è stata costruita, non solo porrà una serie di problemi, ma - soprattutto - ha un profilo di forte iniquità sociale: premia i proprietari con redditi e patrimoni elevati e penalizza le fasce deboli, massimamente l'istituto dei canoni concordati nelle aree ad elevata emergenza abitativa.

i vincoli e le compatibilità di finanza pubblica *pro quota*, una parte di quelle risorse che non sono entrate si scaricheranno in tagli e riduzione di risorse per i Comuni medesimi.

una riduzione significativa dell'imposizione fiscale sui proprietari immobiliari a reddito elevato ed un progressivo indebolimento delle politiche a favore degli inquilini, scaricando così sui Comuni una serie di ulteriori contraddizioni. È dimostrazione di ciò il fatto che avete tagliato il Fondo sociale per l'affitto e che anche quella modesta misura che era stata introdotta per una sorta di intervento a favore delle famiglie numerose è stata completamente cassata.

Certo che possono non applicarla: il problema è che se li avete ridotti alla fame qualcuno cercherà di approfittarne e di usare quell'opportunità. Quindi, siete voi che avete la responsabilità di aver indotto un incremento della pressione fiscale! ministro Calderoli, non è vero che in questa maniera si premino i virtuosi, perché se lei fa tanto riferimento - com'è giusto fare - alla spesa storica e alle sue disarmonie, chi le dice che quei Comuni che non hanno finora abbiano fatto solo perché potevano giovarsi nel tempo di una spesa storica e di trasferimenti più vantaggiosi? Quindi, la beffa è doppia per quei Comuni che sono stati costretti ad usare maggiormente le addizionali e che oggi sono in difficoltà e non hanno strumenti se non quello di tagliare i servizi o di aumentare le tariffe.

Voi l'avete computata estendendo al massimo la base imponibile, pur sapendo che ci sono dei meccanismi che la ridurranno, in termini di gettito. Per cui, di fatto, si scaricherà un'ulteriore pressione, soprattutto sulle seconde e terze abitazioni e, in particolare, sulle attività artigianali, commerciali e dei professionisti: è incontestabile che si determinerà l'aumento della pressione fiscale. Altro che riferimenti a non si sa bene quali responsabilità del passato!

E come fate a dire che così è «vedo, voto, pago»? È un'offesa all'intelligenza e al buonsenso! Propongo almeno una formulazione diversa, signor Ministro: vedo con il satellitare, pago salato voto a prescindere. Così mi convince, perché così in base al decreto, ma non è il principio di beneficio che fonda il rapporto di responsabilità e di controllo tra amministratori e amministrati.

- ci sono Comuni che, in forza della spesa storica, hanno avuto opportunità maggiori e altri che devono scontare delle penalizzazioni; quindi, è un discorso generalizzato.

perché noi ne togliamo due, con questa proposta: l'addizionale IRPEF e la TIA-TARSU. Devo dire che, con quella sventagliata di aumenti di imposizioni che voi determinate con questo provvedimento, l'ICS è una soluzione paradisiaca per i cittadini, oltre che essere coerente con i principi della legge n. 42 del 2009, cioè di beneficio e di relazione di cittadinanza tra cittadini e i loro amministratori.

rinunciare a un po' di propaganda e prendersi un po' di tempo per discutere di queste questioni. Anche la discussione di oggi dimostra che c'erano gli spazi per potere fare una buona proposta nell'interesse della generalità dei Comuni e dei cittadini. Guardate che noi mettiamo mano ad una cosa che dovrebbe avere l'ambizione di una riforma strutturale epocale. In realtà, avete combinato un pasticcio, e noi questo pasticcio non vogliamo condividerlo. Signor Presidente, onorevole Ministro, cari colleghi che resistete a questa maratona, cercherò di acquisire la vostra benevolenza

ho ritenuto opportuno l'intervento in Aula proprio per sottolineare e segnalare - il Ministro ne è consapevole e ne siamo consapevoli tutti - che si tratta di una procedura assolutamente straordinaria, eccezionale, che non può costituire, in quella che è e sarà la giurisprudenza in materia di leggi delegate un precedente tale da

convinzione che tale decreto potesse rappresentare una specie di clava per abbattere il Governo, con ciò dando luogo anche ad un confronto aspro, cosa che non si era verificata per i precedenti decreti, e che mi auguro non si verifichi per i successivi. il caso che si è verificato in Commissione bicamerale è di una parità che si potrebbe definire "contro natura", perché non rappresentava più lo schieramento parlamentare del Senato e della Camera, ma un nuovo un nuovo schieramento dovuto all'impossibilità di sostituire, almeno in quel frangente, i propri componenti. Spero che anche di questo si faccia giustizia e si ritorni alla normalità dell'equilibrio interno della Bicamerale. Detto ciò, signor Presidente, Presidente, occorre affermare con forza che, una volta che il legislatore ha conferito al Governo una delega, quest'ultimo è tenuto a rispettare la delega per i termini, per gli oggetti che devono essere individuati e per i principi e criteri direttivi, che, nel formulare il testo definitivo, il Governo - nell'ambito di quei limiti che ha posto il legislatore delegante - deve avere la

un parere contrario. In realtà, la Commissione bicamerale non ha approvato un parere contrario, che probabilmente avrebbe determinato la necessità dell'attivazione della procedura prevista in via particolare dalla legge delega, la legge n.

conto dell'evoluzione del dibattito e dei contributi dati, sia interni alle procedure fissate dal legislatore, sia provenienti dall'esterno. Questo perché, se il Governo si accorge di aver commesso un errore di natura legislativa, credo credo possa determinarsi in un senso diverso ancorché questo difetto non sia stato sollevato nell'ambito di una formale procedura parlamentare. Mi auguro soprattutto che queste vicende non abbiano a ripetersi su un tema così delicato come il federalismo e che si possa ritrovare quel clima di serenità che mi sembra abbia sempre contrassegnato il percorso relativo all'attuazione dell'articolo 119, sia nella formulazione della legge delega che nei decreti delegati.

La seduta è tolta